Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, se fossimo a scuola l'insegnante mi direbbe che sono ripetitiva. Ma tant'è, siamo alle solite, con i Governi Conte che sembrano caratterizzati dalla ma che invece fa capire quanto sia ampio il *gap* tra l'azione del Governo e la realtà dei gravi problemi del nostro Paese, che richiedono invece interventi urgenti e soluzioni. Nella realtà dei fatti la maggioranza copre con l'ideologia le vere motivazioni del proprio operato; si serve dell'emergenza, in particolare dello stato di emergenza, per garantire la sopravvivenza del Governo, ma non riesce ad assumere poi decisioni nette e coraggiose sulle questioni essenziali, anche perché le diverse componenti non sono d'accordo proprio su nulla. Ad oggi il Governo cosa ha concluso? Alitalia, Ilva, Atlantia, TAV TAV no, MES sì, MES no, tavoli di crisi aziendali irrisolte: sono questioni non affrontate tempestivamente, aggravatesi casomai con la crisi in corso, rimaste irrisolte e divenute veri tormentoni. Le previsioni sono allarmanti: il PIL è previsto in forte calo, *idem* la produzione industriale; i consumi interni sono fermi, mentre il debito pubblico raggiunge quota 158 per Qual è la risposta? Pronte nove milioni di cartelle esattoriali per accertamenti, aumento di bollette, misure non finanziate a sufficienza, tasse non prorogate né tantomeno diminuite. La priorità rimane il lavoro. Secondo la CGIA di Mestre, entro la fine dell'anno saranno persi circa 3,6 milioni di posti di lavoro, ma non ci possiamo stupire; non vi sono investimenti *shock* sulle imprese e il mondo del lavoro continua a essere ingessato quando invece sarebbe opportuno poter creare più possibilità. Anche in questa occasione non sono state accolte le nostre proposte per renderlo più snello e flessibile: dall'abolizione delle causali all'addizionale per le proroghe dei contratti a tempo determinato all'inserimento dei *voucher*, all'introduzione di veri incentivi non solo per le assunzioni, ma anche per il mantenimento dei posti di lavoro. Il problema è che non vi sono progetti né a medio né a lungo termine. La mentalità di questo Governo è di tipo assistenzialista, e non propensa a investire per far girare l'economia e creare PIL. Non si risolvono strutturalmente i problemi dell'occupazione; si aumenta la spesa corrente e il *deficit*, si creano le premesse per il definitivo fallimento di migliaia di imprese: o si programmano interventi strutturali lungimiranti, non limitati a vecchi progetti di opere tirate fuori e rispolverate dai cassetti ministeriali, oppure non ci sarà futuro.

che la misura ancora non parte. Sono mesi che il settore non lavora perché i committenti sono in attesa del superbonus, per poi scoprire che il provvedimento implica pali e paletti e tanta, tanta burocrazia che ne limiterà enormemente la portata. Il Governo Conte basa i suoi progetti futuri sulle risorse provenienti dal *recovery fund*; peccato che l'Esecutivo sia molto indietro sui piani. Intanto, con l'ennesimo annuncio in anteprima, viene lanciato lo stato di emergenza per la crisi sanitaria Covid-19 almeno fino al 31 gennaio prossimo, Bisogna infine sottolineare come questo Governo viva fondamentalmente di annunci, ma se - come capita spesso - gli annunci vengono diffusi prima della promulgazione della norma o del decreto del è fatale, soprattutto in questa fase di emergenza, perché si provocano distorsioni che possono essere anche pesantemente lesive degli equilibri di mercato e controproducenti dal punto di vista sociale, e ciò è molto grave. Anche per questo abbiamo il dovere di continuare a gridare il nostro sdegno per le decisioni scellerate di questo Governo, prese a colpi di DPCM, di decreti-legge, di provvedimenti attuativi, cui si aggiungono - se non se ne fosse abbastanza - anche le circolari dell'Agenzia delle entrate tanti provvedimenti che spesso si spingono oltre all'enorme legiferate - e questo è gravissimo - ma che nella sostanza rivelano l'immobilismo dell'azione del Governo e dove agiscono, invece, fanno danni. caso della decisione di investire circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di banchi, tra cui quelli a rotelle - e vorremmo fare anche un'altra interrogazione per capire il costo reale - per fronteggiare le limitazioni imposte dall'emergenza Covid nella scuola, a differenza del Governo tedesco del Governo tedesco che invece allo scopo ha deciso di investire mezzo miliardo per la digitalizzazione delle scuole. Il risultato è che in troppe scuole italiane - ricordo l'esempio di un istituto professionale di Venezia gli studenti non fanno lezione né a scuola né a casa, perché mancano sia insegnanti che strutture idonee, e non riescono nemmeno a fare la didattica a distanza. Questa è la differenza tra un Governo che interviene efficacemente, guardando in prospettiva anche al futuro, e un Governo, come il nostro, che invece spende male le risorse e fatica a rimediare ai problemi, limitandosi all'ottica del presente. Signor Presidente, intervengo in questa discussione generale sulla fiducia. La posizione che il mio Gruppo esprimerà credo che sia ovvia, ma la specifico a beneficio di chi ci ascolta fuori da quest'Aula: noi naturalmente voteremo contro. Mi limiterò a dare qualche argomento, sia sul metodo che nel merito del perché voteremo contro. Partirò da quella che potrebbe essere la lapide che verrà posta sulla tomba di questo Governo al prossimo appuntamento elettorale: «Avevano annunciato la lotteria degli scontrini, realizzarono la lotteria delle cartelle. Gli elettori riverenti posero». Sì, perché la lotteria degli scontrini è stata posposta al 1° gennaio, mentre il 15 ottobre partiranno 9 milioni di cartelle; un po' alla volta, però, ci ha detto il signor Ministro dell'economia e delle finanze: partiranno con delicatezza e quindi, qualcuno se le troverà nella cassetta della posta, in una situazione economica del Paese che è quella che conosciamo. E lo è anche perché

ad esempio, invece di venire in Assemblea a piangere lacrime di coccodrillo sulle sorti delle attività che chiudono, non si potevano trovare 500 milioni di euro per prorogare fino a fine anno il credito di imposta sugli affitti commerciali? Avrebbe potuto essere una misura che avrebbe consentito a tante piccole attività di provare a resistere fino alla fine dell'anno, nell'attesa che riparta l'economia. Invece no. no. L'atteggiamento di questo Governo è quello che ho già descritto: è l'atteggiamento della lotta contro i kulaki, della lotta ideologica contro la proprietà, in particolare contro la piccola proprietà, perché la grande proprietà, la grande finanza in molte anime di questa maggioranza trova ascolto. Voglio fare un esempio, signor Presidente, che non è tratto dal provvedimento in esame, ma che in qualche modo è l'epitome di questa filosofia di intervento.

All'articolo 6 di questo disegno di legge - pensi che cosa si è inventata questa maggioranza - è previsto che i Comuni censiscano e mappino gli immobili commerciali localizzati nei centri urbani storici inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado degrado urbano causato dal loro inutilizzo, possano modificare in aumento l'aliquota di base dell'IMU fino a tre volte. Non so se mi sono spiegato.

senza precedenti e interventi non risolutivi da parte del Governo fanno chiudere le attività commerciali? di intervento, e cioè di uso del fisco prevalentemente in chiave punitiva, non ci deve stupire: alla fine è la stessa filosofia dell'IRAP, la grande invenzione dell'onorevole Visco che, penalizzando il costo del lavoro, pensava che gli imprenditori si sarebbero spostati sul capitale, sulle macchine e che questo avrebbe fatto aumentare la produttività, sulla base dell'idea, anti imprenditoriale e anticapitalista, che l'imprenditore è un pigro, un ricco, un padrone, un parassita, che tendenzialmente campa di rendita. Questi imprenditori ci saranno anche, per carità: ogni cesto ha delle mele marce - tranne questa maggioranza beninteso - e, quindi, può anche essere che sia così. Gli imprenditori che vedo io si svegliano ogni mattina

una crisi di domanda senza precedenti (già evocata, ma ricordiamola) e - *last but not least*, per esprimerci come parlano al

parla di tutto affinché non si possa approfondire niente e che si tramuta poi, fatalmente, nelle Commissioni - perdonatemi il neologismo, spero che non venga censurato dalla Presidenza -, in un marchettificio su cui poi si abbatte la mannaia della Ragioneria generale dello Stato,

nel tessuto produttivo e per le famiglie in difficoltà, qui c'è una maggiore attenzione alla ripartenza economica, anche se devo dire non risolutiva. Penso soprattutto alla norma che esonera dal versamento contributi previdenziali quelle imprese che rinunciano alla cassa integrazione, ma vanno in questa direzione anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la moratoria su prestiti e mutui, il Fondo di sostegno alle realtà che partecipano ai progetti di interesse europeo. Con il provvedimento in esame si è cercato un punto di equilibrio tra rilancio e assistenza, che comunque non deve mancare perché ci sono settori e categorie ancora in grandissima difficoltà. quindi, la riprogrammazione delle scadenze fiscali, così come gli aiuti a quelle categorie che non ne avevano beneficiato, come gli stagionali del settore turistico e termale. al turismo, è importante la norma sui crediti di imposta per gli affitti, anche se il timore è che tutto questo non sarà sufficiente. Senza essere catastrofisti, l'aumento dei casi di contagio getta una pesante ombra sulla stagione invernale, per non parlare delle città d'arte che, senza il turismo straniero, sono praticamente al collasso.

aiutare e venire incontro a quelle aziende e agli occupati in quei settori se veramente questa pandemia non ci lascerà liberi. Presidente, su un provvedimento che pesa 25 miliardi di euro, la quota destinata al lavoro parlamentare è stata di appena 250 milioni di euro. Ancora una volta devo e voglio esprimere il mio rammarico per il fatto che Commissioni venga lasciato così poco margine di manovra. Eppure, precedenti provvedimenti hanno dimostrato che il Parlamento è riuscito a rendere migliori le misure di rado in uno spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizioni, com'è accaduto anche in questa circostanza. In Commissione ci siamo fatti carico delle situazioni di fragilità, come quelle dei lavoratori immunodepressi, dei malati oncologici, dei territori colpiti dal sisma, del turismo e del settore termale, degli ambulanti. i territori che rappresentiamo, purtroppo non si riesce ancora a scrivere una parola fine sul rinnovo della concessione della A22. L'Autobrennero è un'arteria di strategica importanza per tutto il Paese,

Grazie, Per concludere, Presidente, oggi licenziamo il provvedimento al nostro esame sapendo che dai prossimi giorni ci attenderà il lavoro sulla legge di bilancio e quello sul *recovery fund*. Senza voler apparire retorici, nei prossimi mesi si deciderà il futuro del Paese. Occorre uscire dalla bulimia delle troppe proposte per mettere in campo un percorso che coinvolga attivamente anche le autonomie territoriali,

e chi vuole investire. Qui non è tanto importante che si opti per il modello tedesco o per quello della riduzione delle aliquote, quanto il fatto che tutti i cittadini possano finalmente sapere cosa pagano, quando pagano e perché pagano. e oggi col MES l'Italia può davvero dare vita alla più grande riforma che abbia mai conosciuto dai tempi dell'introduzione del Servizio sanitario

quel giorno prima o poi arriverà. Solo con la crescita si riduce il debito di un Paese; solo con la crescita si creano posti di lavoro, come purtroppo ci insegna anche il fallimento del reddito di cittadinanza come politica attiva per il lavoro: una crescita nuova comunque, una crescita indirizzata tutta sulla sostenibilità; una crescita che garantirà per arrivarci ci vuole tutto il protagonismo del sistema produttivo. È su questo che dobbiamo continuare a lavorare è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.

approvati per tamponare la grave crisi economica, sanitaria e sociale che il Covid ha comportato per il nostro Paese. Sono dieci mesi di interventi, 100 miliardi di nuovo indebitamento netto, 210 miliardi di saldo netto da finanziare. Sono numeri capaci di raccontare nella loro efficacia tutta la drammaticità e anche la straordinarietà del momento che stiamo vivendo.

un percorso che ci veda realmente percorrere la via della rinascita e della resilienza del nostro Paese. Quindi in questa Aula oggi, con l'approvazione del decreto agosto, va detto molto chiaramente che crescere, ritornare a crescere, è non una scelta, ma un obbligo imprescindibile per il nostro Paese. Siamo in un momento difficile e rischiamo moltissimo. Per avere parametri di finanza pubblica buoni e, quindi, lavoro e benessere diffuso, serve per prima cosa evitare,

Un'altra questione prioritaria è iniziare a lavorare con massima serietà per ottenere le risorse del *recovery fund*, del piano Next generation EU. gli obiettivi, li abbiamo sentiti decantare in moltissime Aule, in questa sede, in Commissione e nelle varie Commissioni bicamerali. È chiaro che noi vogliamo costruire un Paese innovativo, dinamico, *green*, socialmente integrato e paritario.

Giovedì approveremo le linee guida sul *recovery fund* e, entro aprile, approveremo il Piano nazionale di ripresa e resilienza Naturalmente e necessariamente dovremo approvarlo a gennaio, non ad aprile, in modo tale da essere il prima possibile nelle condizioni di ricevere il primo acconto dall'Europa. Il *recovery plan* e il PNRR sono un patto sociale e politico; certo, sono la decisione di dove, come e quando investire le risorse: è fondamentale e importantissimo. Si può dire per il nostro Parlamento e la nostra democrazia, ma sono soprattutto un bivio: decidere di avere una nuova generazione europea in Italia, oppure lasciarci scivolare nell'inedia, nelle scaramucce politiche quotidiane, negli interessi di parte o nella lentezza di alcune burocrazie. Quello che affronteremo giovedì è quindi non un fatto cartaceo, ma un fatto esistenziale. decreto agosto, pur avendo investito 25 miliardi, non è stato propriamente un passaggio esistenziale; un passaggio sicuramente importante, ma una misura calata ancora nella fase di emergenza, molto ricca di aiuti necessari e indispensabili in questa fase. Si tratta però pur sempre di aiuti. Abbiamo visto molte proroghe di misure adottate nel cura Italia e nel decreto rilancio; molta cassa integrazione e ancora indennità, *bonus,* giustamente diritti per lo *smart working*, risposte agli eventi calamitosi (dalle gelate alle alluvioni) e poi ampliamenti dell'ambito soggettivo per accedere alle garanzie del Fondo garanzia PMI; ampliamenti dell'ambito soggettivo per accedere al *bonus* ristorazioni;

non si vede nulla di decisivo per la rinascita, la resilienza e la ripartenza del nostro Paese. Dobbiamo ancora accogliere moltissime delle istanze del mondo produttivo, che chiede di potersi modernizzare, di poter pagare, giustamente, le tasse, ma incentivando tutti i fattori produttivi, di potersi aggregare e di diventare più competitivo, di essere messo nelle condizioni di trainare questo Paese fuori dalla difficoltà. Ancora non abbiamo affrontato il nodo del reddito di cittadinanza. È chiaro, ormai, a tutti noi che, così come è stato

del Paese. In questa fase dobbiamo dirci che servono dei prerequisiti, un cronoprogramma di lavoro, delle linee strategiche per evitare di perdersi ancora in singole richieste in singoli interventi di aiuto. Sarà anche una politica faticosa, sarà anche una politica poco popolare, quella seria, ma in questo momento non abbiamo moltissime alternative. Nel momento della grande responsabilità di traghettare il Paese fuori da questa meglio farlo con una sorta di unità nazionale, dove tutti sono chiamati a responsabilità. Sicuramente la maggioranza deve cambiare atteggiamento e deve averne uno nuovo per rialfabetizzare il Paese. Abbiamo fatto molto sulla coesione sociale e territoriale, ma sulla rialfabetizzazione del Paese ancora non abbastanza, come sulle competenze digitali e infrastrutturali e sul piano del dissesto idrogeologico. Mi sembra che le immagini drammatiche di questi giorni dicano molto sui ritardi che dobbiamo colmare: infrastrutture, ponti, porti e metropolitane. Mi pare che in questo momento, e lo dico unendomi a chi lo ha chiesto con forza, serva un punto politico di maggioranza: un programma chiaro, strategico, e maggiori competenze. Maggiori competenze, perché, quando i problemi da risolvere sono difficili, servono maggiore competenze e soggettivo coraggio nell'affrontare le decisioni, anche impopolari. tutto questo non è chiesto solo alla politica, ma è chiesto a tutte le classi dirigenti, ai corpi intermedi (da Confindustria alla CGIL), che ci stanno stimolando da questo punto di vista, e anche ai dirigenti, pubblici e privati. Qui è in gioco il futuro di tutti, anche di quelli che, fino ad oggi, sono stati i più garantiti. Quindi, questo messaggio deve entrare nel circuito mentale di tutti. Tutti, perciò, devono mettersi in gioco, studiando di più, facendo più fatica e anche cercando di porsi nella prospettiva di una politica dei fatti. E i fatti non sono compatibili ai rinvii. Talvolta i *dossier* sono complessi, le decisioni anche. Sono difficili da assumere, ma sono inevitabili. Allora, in questo momento, la decisione di affrontare lo strumento dell'ammortizzatore sociale unico diventa imprescindibile. Abbiamo visto che sono serviti quattro decreti-legge per colmare tutte le lacune degli attuali strumenti di garanzia, che non sono compatibili né con l'emergenza né con un Paese come quello che vogliamo costruire. Dobbiamo decidere sul MES. È solo una decisione logica, non è una provocazione politica.

partire con le infrastrutture e non tener fermi i *dossier* di investimento. Visto che lo hanno citato gli altri colleghi, cito uno dei principali investimenti, che è l'autostrada del Brennero, la principale infrastruttura di collegamento tra Italia ed Europa. Questo decreto-legge poteva trovare delle soluzioni, ma non ha voluto trovarle. Era piuttosto semplice trovarle, perché, come ha detto il collega Steger, questa è già una *in house*, dotata di capacità di investimento importante e indispensabile in questa fase, e basta solo lasciarla proseguire nella virtuosa efficacia della sua azione. Invece, si è voluto insistere su una proposta *ad personam*, in deroga al codice civile, che, giustamente, la Presidenza del Senato ha dichiarato improponibile. con un pensiero di De Gasperi, che ci unisce in una fase di ricostruzione: «Bisogna dire, francamente, che gli organi dello Stato si sentono insufficienti se non si sentono integrati dalla collaborazione delle categorie interessate, da un dinamismo di adesioni e concorsi, che suppone un alto grado di solidarietà sociale. Non c'è nessuna formula magica, nessun Governo, nessuna organizzazione l'ha mai trovata, o meglio la formula c'è, ma è assai complessa: è la solidarietà, è il senso morale, è la coscienza civica al di sopra degli odi di fazione, dell'egoismo di classe, delle manovre politiche, di tutte queste cose piccole e deteriori in confronto alla salvezza del popolo italiano». A questa prospettiva Italia Viva vota sì.

dell'illustrazione della relazione di minoranza che mi è stata concessa, il ringraziamento a tutta la Commissione per questo lavoro fatto e per averci quantomeno, per la prima volta, consentito di arrivare a valutare approfonditamente le proposte che sono arrivate sul tavolo della Commissione, che per la prima volta hanno visto le relazioni tecniche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Oltre a questo ringraziamento, volevo anche denunciare, Presidente, un comportamento secondo me e secondo il mio Gruppo scorretto da parte di questo Governo e di questa maggioranza, che pensava - voglio usare termini equilibrati - di condizionare le minoranze, concedendo loro 25 milioni di euro su un decreto di 25 miliardi di euro sotto forma di proposte da inserire attraverso emendamenti a questo decreto che oggi è in discussione. Su queste elargizioni, il Gruppo Fratelli d'Italia aveva l'opportunità di avanzare richieste per cinque milioni di euro, ma anche se fossero stati cinque miliardi di euro, li avremmo chiaramente rispediti al mittente, perché non ci siamo mai prestati a questi giochi da manuale Cencelli sulla pelle degli italiani. invece, in questi mesi ha avanzato migliaia di proposte e ha chiesto al Governo di valutarle entrando nel merito delle stesse. Questa era la collaborazione che chiedevamo non possiamo e non accetteremo mai che ci vengano concessi cinque milioni di euro come fosse un prezzo da pagare per poter dire che collaborazione e dialogo ci siano stati all'interno della Commissione prima e di questa Assemblea dopo. Noi non siamo in vendita, il nostro onore e la nostra dignità non hanno un prezzo che si possa pagare. Quindi, Presidente, siamo ancora una volta qui a recitare una commedia. Il Governo, come abbiamo sempre detto e denunciato, non ci ascolta, decide da solo e non sente il Paese e questo è un grave fatto che non ha precedenti nel nostro Paese. Continuate a chiamarci a ratificare scelte già prese, senza un minimo di collaborazione, senza un minimo di confronto. Voi pensate

e a cui voi avete dato, attraverso questa misura approvata con il decreto rilancio, un solo anno di tempo per dispiegare la sua efficacia, sapendo che poco più di un anno non basterà nemmeno per poter ottenere i titoli autorizzativi che tutti coloro i quali avranno bisogno di questa misura dovranno richiedere ai propri enti locali.

aspettandovi, come vi siete impegnati, sulla legge di bilancio per vedere se ci saranno le condizioni per rendere strutturale tale norma, tale norma, che - voglio ribadirlo - prevede una delle pochissime misure, in un contesto di 100 miliardi che avete sperperato, che può dare una speranza di sviluppo vero al nostro Paese. Su questo vi sfideremo - ripeto - nella manovra di bilancio per capire se manterrete gli impegni che vi siete presi attraverso l'approvazione di questo ordine al giorno presentato dal Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia. Purtroppo, il cosiddetto decreto-legge agosto segue la stessa logica e la stessa scia dei precedenti decreti: tanto assistenzialismo e zero misure in grado di mettere le basi per uno sviluppo concreto, serio e reale del nostro Paese. Paese. Come ho detto prima, avete sperperato 100 miliardi di euro, che - badate bene - non sono miliardi dati a fondo perduto, bensì un debito che lascerete in eredità alle future generazioni.

delle occasioni mancate perché, come ho sempre detto, manca una spinta per la ripartenza. Purtroppo, dobbiamo constatare di nuovo che non è stato fatto nulla nemmeno in questo provvedimento, nel quale speravamo che, essendo l'ultimo di alcuni decreti emergenziali, ci fosse una visione politica per lo sviluppo del Paese. Voi continuate ad operare e a vivere tamponando esclusivamente l'emergenza, che in parte può essere certamente un fatto legittimo, ma fuori da quest'Aula c'è un Paese che chiede di essere messo nella condizione di camminare con le proprie gambe. A questo Paese voi consegnate l'ennesimo provvedimento infarcito di burocrazia e nemmeno l'ultimo decreto semplificazione ha dato la possibilità di risolvere queste problematiche. La vostra regola è sempre stata quella di dire: rinviamo al prossimo decreto. Oggi con questo provvedimento ci avete detto che rinvieremo ancora e che tutto sarà fatto con i fondi del *recovery fund* (209 miliardi).

voi avete avuto il coraggio - perché non era nel testo base - di approvare un emendamento qualche sera fa con il favore delle tenebre, mentre nella legge di bilancio non vi era stata concessa questa possibilità, per approvare un emendamento di 900.000 euro legato alla Casa internazionale delle donne di Roma. Questa è una cosa che non si può sentire; avete fatto approvare questo emendamento per evitare lo sfratto ad un'associazione nella città di Roma Capitale. Mi dovete spiegare cosa c'entra la Casa delle donne di Roma con un decreto emergenziale. Non capisco perché nessuno denuncia questi fatti, a parte noi che facciamo parte dell'opposizione. Collega Manca, i 20 milioni di euro per le consulenze al ministro Franceschini cosa c'entrano con questo decreto? Il riassetto del gruppo SACE, le consulenze del ministro Gualtieri, le assunzioni all'arsenale militare di Taranto, cosa c'entrano con questo decreto emergenziale, collega Manca? A queste domande non abbiamo trovato risposte. Abbiamo presentato emendamenti chiari, precisi e puntuali per eliminare alla radice queste

tutte caratteristiche che evidentemente sono mancate a questo Governo e a questa maggioranza ed è per tali motivi che Fratelli d'Italia non voterà mai e poi mai la fiducia a questo Governo.

dai relatori e dai membri della Commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione. È stato un lavoro assai importante per un decreto-legge molti hanno detto e io voglio ricordare, è praticamente il quarto della serie dei provvedimenti di emergenza. Ho sentito qui ancora una volta le critiche su questo aspetto, ma credo fosse responsabilità di tutti tutti intervenire per la proroga di alcune misure - penso alla vicenda della cassa integrazione, agli sgravi contributivi, alla proroga della NASPI (nuova

con cui è stata sanata l'ingiustizia che si era venuta a creare per la mancata proroga delle tutele nei confronti dei lavoratori fragili e degli immunodepressi È stato un intervento importante che, come i relatori sanno, è stato centrale anche nella ripartizione delle risorse. A questo si aggiunge

poi l'intervento sul turismo, sulle terme. Sappiamo perfettamente che il comparto del turismo è stato tra quelli più provati e probabilmente dovrà ancora affrontare molte difficoltà, ma abbiamo voluto concentrarci anche qui su una serie di misure assolutamente importanti per le imprese turistiche, con la proroga, anche della cassa integrazione per i lavoratori del turismo, il rafforzamento delle indennità, la *tax credit* affitti, la sospensione

continuare. Penso ad alcune misure importanti per quanto riguarda il sistema sanitario e all'approvazione di alcuni emendamenti tra

temi, che pure sono stati inseriti, ad esempio il settore ambientale. Finalmente, dopo tanto tempo e dopo che all'unanimità la Commissione ambientali aveva spinto per l'approvazione del disegno di legge contenente questa norma, è stata eliminata un'anomalia tutta italiana, che stabiliva una percentuale non superabile per l'utilizzo della materia prima seconda, ad

Avete ascoltato spesso i miei interventi al riguardo. Certo che abbiamo bisogno di una visione, di una progettualità ampia, di una strategia e di concentrarci sulle priorità: questi sono stati decreti fondamentali per tamponare l'emergenza e oggi siamo tutti alla prova per dare un futuro a questo Paese, ricordando quali sono le sue priorità. Si è parlato molto di dissesto: certo che servono altre risorse, ma anche quelle che ci sono dobbiamo trovare il modo di

è arrivato il momento di cambiare strada e di fare in modo che, quando si discute, si approvino le norme e ci si assuma la responsabilità di quello che si vota,

il decreto che ci apprestiamo a convertire contiene misure importanti per il sostegno al reddito e alla ripresa dell'attività economica delle persone e delle imprese più colpite dalla crisi economica e sociale innescata dalla pandemia. È per questo che quello del Partito Democratico è un sì convinto a un provvedimento che cerca di non lasciare nessuno da solo di fronte alla fatica di non restare schiacciato sotto gli effetti drammatici della crisi. Tuttavia, la soddisfazione di chiudere con la conversione di questo decreto-legge non deve farci perdere di vista la prospettiva in cui dobbiamo inserirlo e la sfida enorme che ancora abbiamo di fronte, ossia quella di non lasciare nessuno da solo nella fatica del cambiamento che ci attende. esame, com'è stato ricordato, è l'ultimo di una serie di interventi importanti, tanto sul piano legislativo quanto su quello finanziario, per dare garanzia del reddito ai lavoratori e liquidità alle imprese e investire sui servizi pubblici di fronte all'emergenza Covid, a partire da sanità e scuola. Adesso serve però una nuova fase: dobbiamo chiudere quella emergenziale, fatta di interventi giustamente ispirati a una logica risarcitoria, cioè volti a risarcire le persone e le imprese per i costi della crisi, e aprirne una progettuale, che metta al centro una crescita sostenuta e sostenibile e la giustizia sociale. partendo da quest'esigenza, voglio ricordare alcune novità di questo decreto-legge, che è vero che si muove ancora in una logica emergenziale e risarcitoria, ma contiene alcuni semi che, se ben interpretati, ci possono aiutare per le sfide che ci attendono. Sul lavoro, rinnoviamo la cassa integrazione d'emergenza per diciotto settimane, nove delle quali senza costi aggiuntivi per le imprese e nove con costi graduati sul calo di attività: per la serie - se interpretiamo bene il messaggio - che non si può stare fermi, stiamo per uscire dalla terapia intensiva del *welfare* e lo Stato c'è, ma si deve tornare a progettare come creare lavoro. Per aiutare la creazione di lavoro, il decreto-legge introduce nuove forme di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato, gli stagionali e le aziende che smettono di usare la cassa integrazione: per la serie - di nuovo, se interpretiamo bene il messaggio - che ora è il momento di misure temporanee, che aiutino chi può tornare a creare lavoro in una congiuntura ancora molto difficile, ma in attesa di un intervento strutturale sul costo del lavoro, sul *welfare* e sulla formazione, che non possiamo rinviare oltre. Nel decreto-legge c'è anche la proroga di due mesi per NASPI e Dis-Coll per i disoccupati e la proroga delle indennità Covid per i soggetti deboli senza altri ammortizzatori sociali, così come c'è un nuovo e importante investimento finanziario sul fondo per le nuove competenze, per mettere al centro dei processi di trasformazione aziendale la formazione e la contrattazione territoriale e aziendale. Per la serie, di nuovo, se interpretiamo bene il messaggio: investiamo su competenza e qualità del lavoro, in attesa di una riforma complessiva e universalistica del *welfare*, preoccupandoci già adesso di finanziare una formazione che non sia la scusa per dare altri sussidi mascherati, ma un investimento di qualità e certificato sulle nuove competenze che servono ai lavoratori. C'è inoltre un intervento importante, fortemente rafforzato nel passaggio parlamentare su richiesta di molti Gruppi, a favore dei lavoratori fragili, immunodepressi, malati oncologici e categorie a rischio di fronte alla pandemia. Ci sono interventi a favore delle imprese e dei professionisti più in difficoltà, con il rafforzamento dei crediti di imposta per il settore turistico e termale, l'esenzione della seconda rata IMU per turismo e spettacolo e il rinvio dei pagamenti per i soggetti ISA in difficoltà. C'è un ordine del giorno, firmato da tutti i Gruppi di maggioranza, che impegna il Governo ad aprire subito un confronto con le Regioni per il riordino e la messa a punto della riforma Un altro seme da raccogliere da questo passaggio parlamentare è il metodo seguito in Commissione bilancio, sotto la guida attenta dei relatori, i colleghi Manca ed Errani, e del presidente Pesco, che ha permesso, più di tante parole sulla centralità del Parlamento, di fare il massimo per migliorare il provvedimento nella situazione data, coinvolgendo anche le opposizioni, che dobbiamo ringraziare per lo spirito costruttivo mostrato in Commissione, pur nella giusta e sacrosanta distinzione dei ruoli. E questo nonostante la sbavatura di ieri, che ha visto saltare alcuni interventi utili, già discussi e votati dalla Commissione; una sbavatura di metodo che deve spingerci a porci qualche domanda e a trovare anche qualche risposta per il prosieguo dei nostri lavori. Detto questo, un minuto dopo la conversione del decreto-legge Governo e maggioranza devono chiedersi come far germogliare questi semi, per passare da una fase emergenziale a una fase progettuale. L'Italia ha un compito enorme, perché, così come ha fatto da apripista in Europa nella gestione dell'emergenza sanitaria, può giocare un ruolo da apripista su un uso progettuale delle risorse che mobiliteremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dove progettuale non sta per sommatoria di mille progetti e di mille rivoli in cui si disperdono le risorse, ma per capacità di mettere in campo un progetto e una visione. Per farlo serve la consapevolezza che i soldi sono importanti, ma non bastano. Per ogni euro che spenderemo dovremo mettere in campo un'idea: un euro, un'idea. Se investiamo un euro sull'edilizia scolastica - e dobbiamo mettercene tanti - dobbiamo metterci una nuova idea di scuola, che ripensi gli spazi e i tempi per aprirsi a territorio e terzo settore, a nuove attività, per farsi comunità educante, combattere la povertà educativa e favorire la mobilità sociale. Se investiamo un euro sulla sanità - e dobbiamo mettercene tanti, usando tutte le linee di finanziamento disponibili - dobbiamo metterci una nuova idea di sanità, per raggiungere la vita delle persone, soprattutto quelle più fragili, con una forte rete di servizi territoriali, non solo ospedalieri (lo ricordava ieri la collega Boldrini) e investendo sulla telemedicina. Se investiamo un euro sul sostegno per le famiglie con figli a carico - e dobbiamo mettercene tanti con la riforma dell'assegno unico - dobbiamo metterci una nuova idea di condivisione della scelta di fare figli all'interno della coppia; non una scelta che le donne da sole devono conciliare con il lavoro, ma una scelta che devono condividere. E allora parliamo di congedi di paternità obbligatori, di *part-time* di coppia agevolato; mettiamoci un'idea di condivisione per rafforzare la libertà di tutti, uomini e donne. Se investiamo un euro sulla garanzia del reddito per chi è in difficoltà - e dobbiamo anche qui in mettercene tanti mettiamoci una nuova idea di *welfare*, un *welfare* universalistico che aiuti tutti, dipendenti e autonomi, poveri e disoccupati, ma con strumenti diversi e con servizi integrati di formazione permanente. Concludo sui destinatari degli interventi, che devono essere sempre più progettuali e non emergenziali; sull'obiettivo che dobbiamo tenere presente quando disegneremo la nuova fase. C'è senza dubbio la transizione digitale ed ecologica da mettere al centro degli investimenti pubblici e privati, come è stato ricordato nella discussione, ma ci sono anche i grandi volani di crescita inclusiva che dobbiamo sapere individuare nel mondo del lavoro; di nuovo, in tutto il mondo del lavoro, dipendente, autonomo e imprenditoriale. Questi volani sono anzitutto due: il lavoro dei giovani e delle donne. Dobbiamo smetterla di parlare di giovani e donne nei nostri convegni per iniziare a metterli al centro dei nostri provvedimenti di spesa e delle nostre riforme. A livello internazionale è partito un appello, *half of it*, ripreso in Italia come il giusto mezzo da una rete di associazioni e personalità per far sì che metà dei fondi dell'Unione europea raggiungano il lavoro e le opportunità delle donne. Non limitiamoci a firmare quell'appello, ma progettiamo politicamente come metterlo in pratica, chiamando a raccolta tutti gli attori sociali e istituzionali intorno a un piano nazionale per l'occupazione femminile e dotandoci di strumenti conoscitivi per valutare l'impatto di genere di ogni misura, come chiede anche un parere approvato dalla Commissione lavoro del Senato, perché il giusto mezzo richiede la giusta attenzione alla valutazione e all'impatto di genere. concludo davvero dicendo che, di fronte a un nemico terribile e visibile, il virus, la maggioranza e il Governo hanno saputo fare anche scelte difficili. Adesso, di fronte a un nemico altrettanto terribile ma meno visibile, come il declino economico e sociale del nostro Paese, servono scelte altrettanto difficili, ma soprattutto servono scelte. Scelte rispetto alle quali non saremo misurati contando i «mi piace» su Facebook domani, ma pesando i giudizi sulla nostra capacità di promuovere la crescita economica e la giustizia sociale dopodomani. Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, innanzi tutto mi sia permesso di ringraziare i colleghi della 5a Commissione, i relatori Errani, Manca, Calandrini per l'opposizione, e i rappresentanti del Governo che si sono avvicendati in Commissione (i viceministri

credo sia fondamentale, in un momento come questo per il Paese, al di là del ruolo di maggioranza e opposizione, affrontare le questioni, anche e certamente con idee diverse rispetto alla visione complessiva, ma

il punto base per affrontare un momento come quello attuale. Stamattina abbiamo avuto la notizia del

è ancora imperante a livello nazionale; manca quel *boom* del terzo trimestre, che invece il ministro Gualtieri ci aveva annunciato qualche mese fa (e questa è una critica che vogliamo esprimere); il crollo del turismo incombe. Ci poniamo continuiamo con un meccanismo assistenziale o vogliamo seriamente tentare delle scelte (nessuno ha la certezza sulle azioni che dobbiamo intraprendere) per indirizzare il cambiamento? C'è troppa frammentazione, troppi *bonus*,

Il tema è: qual è la visione del futuro? Viene la battuta, fatta anche dai miei colleghi questa mattina: sono i 9 milioni di cartelle esattoriali che Ci rendiamo conto che lo Stato deve attivarsi per il recupero, però vorrei anche ricordare che sono sei mesi che questa opposizione vi sollecita a fare un piano ragionevole, a non continuare con l'acqua alla gola a prorogare di otto giorni in otto giorni. *(Applausi)*. Era questa la questione. Devono protestare e minacciare lo sciopero alcuni dottori commercialisti, per arrivare poi a ottenere una proroga di un mese, con relativi interessi

si riferisce a un milione di lavoratori in meno. Ci rendiamo conto che il reddito di cittadinanza non funziona o, almeno, non funziona per la parte relativa alla Ha funzionato a livello assistenziale, lo ammettiamo, perché in qualche modo ha rappresentato quel *recovery money* che avevamo richiamato sei mesi fa; però c'è ancora un'ottusità nel non volere un po' di flessibilità nel mercato del lavoro. I *voucher* sono un meccanismo per regolare e per immettersi nel mercato del lavoro: è politica attiva del lavoro. crescendo il lavoro in nero. Noi vogliamo essere complici di tutto ciò e poi denunciarlo? È questa la questione. Noi siamo per risolvere. L'eccesso di ideologismo fa dei danni. Vi è poi la questione della liquidità, in qualche modo tamponata; ciononostante, ad ogni provvedimento dobbiamo intervenire sul fondo di garanzia o correggendo una parte della platea.

Parlamento. Noi denunciamo che non ci fornite un disegno complessivo. Da parte della maggioranza non c'è un disegno complessivo. Chi vi parla è a favore dell'utilizzo del MES: ci volete dire se l'intervento nella sanità verrà fatto utilizzando dei tassi vantaggiosi, con meno vincoli rispetto al *recovery fund* che tutti propagandiamo? *(Applausi)*. Vogliamo cogliere l'occasione per modernizzare il nostro sistema sanitario e creare tutte quelle stabilizzazioni che sono necessarie

che dia sicurezza agli italiani e permetta il coraggio degli investimenti. Noi dobbiamo far crescere la parte pubblica con le infrastrutture e la parte privata con gli investimenti privati e affrontando la sfida che ognuno di noi ha,

i membri del Governo che velocemente sono stati disponibili, nonostante fossero molto presi dal fare riunioni per cercare di trovare equilibri in una maggioranza che

Ci siamo ridotti, anche questa volta, di fronte a un provvedimento così corposo, a votare gli emendamenti di notte perché non si riusciva a trovare la quadra sugli argomenti sui quali si era convenuto di

perché la questione si risolvesse. Alla fine la maggioranza è uscita con un ordine del giorno piuttosto ridicolo. Però questa era un tema da affrontare. Sulla riforma delle camere di commercio noi siamo sempre stati contrari, ma abbiamo presentato più di un emendamento in di buon senso: le camere di commercio che hanno bilanci in pareggio e sono virtuose possono non accorparsi, perché secondo noi l'autonomia vuol dire responsabilità e lavoro ben fatto, è stato spazzato via tutto. Vi assicuro che l'atmosfera era davvero molto pesante, ma noi siamo rimasti e abbiamo accettato di lavorare di notte, perché nel provvedimento

più volte abbiamo detto che siamo responsabili, usiamo il buon senso e cerchiamo di aiutare, ma il tempo è finito, perché una volta, due volte, tre volte va bene, ma avete dimostrato nei nostri confronti di opporre blocco ideologico, per cui tutte le proposte di buon senso vengono bocciate in modo aprioristico. Parlo per esempio dei *voucher* nel turismo e in agricoltura.

Poi ancora, le proposte sulla cedolare secca e la questione ormai annosa dei precari storici: come si può non pensare di utilizzare utilizzare gli insegnanti che lavorano già nelle scuole da tanti anni per arginare un'emergenza come quella del sostegno? Come si possono

E ancora, la nostra proposta di estensione della decontribuzione al Sud a tutto il territorio nazionale. Per carità,

e non ciò va assolutamente bene. La preoccupazione è che l'indebitamento è cresciuto ancora una volta, anche con i 25 miliardi di euro che sono stati messi in questo provvedimento. Va bene, tutti avremmo voluto già negli anni scorsi aumentare il debito per una manovra espansiva, ma non era possibile. L'emergenza Covid lo ha reso possibile, direi la tragedia Covid perché non dimentichiamo tutti i morti che ci sono stati e quanto tutti dobbiamo attrezzarci per arginare un'eventuale seconda ondata.

possano generare nuove economie. Non possiamo aspettare però il 2022 e il 2023 perché l'emergenza di chi deve dare la cena ai propri figli, pagare l'affitto o vivere dignitosamente (al minimo, ma vivere) bisogna affrontarla adesso. La cassa integrazione però finirà e quindi come faremo dobbiamo aiutare coloro che danno il lavoro e accettano di rischiare per esso.

per chi è affetto da problemi e disturbi dello spettro autistico. L'abbiamo potuto fare solamente per il 2020, però abbiamo preso

l'educativa scolastica a questi bambini e a questi ragazzi. Il numero sta aumentando incredibilmente e non si possono lasciare sole le famiglie. Un'altra proposta che abbiamo dovuto

a 50.000 ragazzi - che era il numero iniziale - di partire con uno strumento che ha dimostrato tutta la sua efficacia?

ci credete neanche voi ed è pazzesco. I colleghi hanno parlato poi di difficoltà

dobbiamo acquisire un'efficienza senza la quale tutto quello che stiamo facendo non prenderà poi corpo. È un problema gigantesco che ci dobbiamo porre.

che il tempo è finito e anche alla luce di quello che è successo nel corso della trattazione del decreto, non ci saranno più buon senso e comprensione. Utilizzeremo tutti gli strumenti che il Regolamento del Senato ci offre e contiene per fare un'opposizione dura. Probabilmente capirete solo questo, probabilmente in questo caso, se noi avessimo chiesto di votare puntualmente e di fare le cose

membri del Governo, colleghi, oggi siamo chiamati ad esprimerci sul decreto legge 14 agosto n. 104, un provvedimento che, che come altri che lo hanno preceduto, ha preso corpo dopo lo *shock* pandemico e a questo *shock* cerca di porre rimedi immediati intervenendo a beneficio di numerosi settori economici. Colgo anche l'occasione per ringraziare il Presidente della Commissione bilancio e tutti i componenti della Commissione stessa. In diversi casi si tratta di settori che, voglio ricordare, non godevano di ottima salute già prima del *lockdown* che soffrivano ancora per gli effetti delle grandi crisi del 2008 e del 2012. Le misure messe in campo con questo decreto non sono solo di protezione, ma puntano al rilancio dell'economia e a corroborare l'azione di ripresa delle imprese colpite dalle conseguenze negative dell'epidemia. Il provvedimento mette in campo 25 miliardi che portano a 100 miliardi il volume totale delle risorse stanziate fra decreto cura Italia, decreto rilancio e, appunto, decreto agosto. Polemiche strumentali a parte, con onestà intellettuale tutti dobbiamo riconoscere che si tratta di risorse molto ingenti, a riprova di come il Governo e il Parlamento abbiano profuso uno straordinario sforzo, sia qualitativo che quantitativo, per combinare misure di protezione ma anche misure prospettiche. Purtroppo, tra i settori economici maggiormente colpiti c'è il turismo. Ed è proprio per questo settore che il decreto-legge prevede un fondo per la filiera della ristorazione. Infatti, gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato, da marzo a giugno 2020, di almeno il 25 per cento... *(brusio)*. PRESIDENTE. Per cortesia,

potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Ma c'è anche un contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, in favore degli esercenti che abbiano registrato, a giugno 2020, un calo del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019, un credito di imposta del 60 per cento del canone di locazione, *leasing* o concessione e l'esonero del pagamento della seconda rata dell'IMU del 2020 per alcune categorie di immobili e di strutture turistico-ricettive. È un provvedimento che pone attenzione anche al mondo dello *sport*, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni nei confronti di leghe, società società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. Viene a loro riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati. È stato riconosciuto un sussidio di 600 euro per i lavoratori dello stesso mondo dello sport. Come dicevo, in perfetta linea di continuità con il decreto cura Italia e con il decreto rilancio, anche nel decreto agosto ci sono misure di prospettiva: si è provveduto al rifinanziamento di alcuni strumenti come i contratti di sviluppo, il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, il *voucher* per l'innovazione,

(dal 30 settembre 2020, il termine viene esteso al 31 gennaio 2021). Sono state riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, è stato previsto un fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi e un fondo di tre milioni di euro per la formazione di coloro che accudiscono persone bisognose. Il valore simbolico di questa misura è importantissimo, perché dà importanza ad un lavoro tanto essenziale quanto invisibile, appunto quello che consiste nell'accudire persone più in difficoltà e provvedere alla casa. Le nostre case sono anch'esse attraversate dalla rivoluzione tecnologica e dunque la formazione digitale è diventata necessaria per acquisire nuove competenze da aggiungere a quelle tradizionali. Così pure voglio ricordare il fondo di tre milioni di euro per i Comuni siciliani maggiormente coinvolti dalla gestione dei flussi migratori, al fine di fronteggiare in modo concreto il problema degli sbarchi. Colleghi, in attesa delle consistenti somme di denaro in arrivo dall'Unione europea, che ci permetteranno di rilanciare gli investimenti necessari al Paese, oggi ci apprestiamo a licenziare questa misura da 25 miliardi di euro, che darà conforto a numerosi operatori economici e li aiuterà a non soccombere davanti a questa crisi del tutto inattesa. Veniamo da un anno in cui la decretazione d'urgenza ha caratterizzato il lavoro del Governo e di conseguenza del Parlamento. Il decreto agosto ne è l'ultima espressione infatti, ma mi chiedo, oltre ogni polemica e contrapposizione politica: che cosa si sarebbe potuto fare davanti ad un'emergenza così repentina e cangiante come quella da Covid-19?

ebbene, su poco più di 100 articoli, 83 emendamenti sono dell'opposizione. Spero che possiate riflettere su questa fiducia ed essere coerenti con quello che avete detto questa mattina, perché questo Governo ascolta ed interpreta al meglio le esigenze dei cittadini, in un clima di collaborazione

«Se i clienti non mi pagano, nemmeno io posso pagare i miei fornitori e così mi sono cacciato in una spirale da cui non sono più riuscito a riemergere. Sono arrivato ad un bivio: pagare le tasse o dare da mangiare alla mia famiglia. Ho imboccato la seconda strada. Non avevo scelta, cosa avrei dovuto fare?». A parlare è l'artigiano trevigiano di cinquantacinque anni che martedì scorso ha tentato di lanciarsi da una finestra del tribunale di Treviso (fermato dai presenti), dopo avere saputo che la sua casa rischiava il pignoramento per l'azione giudiziaria avviata da quattro suoi creditori. Se volete sapere che cosa significano 9 milioni di cartelle esattoriali, bene, questo è l'esempio. Certo, se un vip è positivo al Covid finisce immediatamente in prima pagina, i contagi sono aggiornati in tempo reale, mentre queste storie finiscono - e lì terminano e lì terminano il loro ciclo - nei giornali locali, perché questa purtroppo è l'Italia che non vedete. Poi ci sono le bollette della luce e del gas, che sono le più vergognose d'Europa per le folli spese spese legate agli oneri di sistema (ma tanto voi siete fermi al decreto agosto e, siccome ad agosto fa caldo e fa buio più tardi, in in fin dei conti vi interessa poco). Penso che siamo arrivati ancora una volta al limite nel vedere che il Parlamento, composto dai rappresentanti del popolo, è tagliato fuori. Mi sono sono quindi miseramente e tristemente rapportato alle storie di questa Italia e mi sono permesso di portarle alla vostra attenzione, dicendo no al vostro decreto-legge.

la dichiarazione che sto per leggere

Qualunque organo collegiale, anche l'assemblea di un condominio, esige che l'ordine del giorno sia dettagliato e siano specificate le questioni da trattare, a pena di nullità, in modo tale che il singolo componente sia messo in condizione di conoscere per deliberare e partecipare quindi in modo attivo e responsabile. Sabato 3 ottobre, alle ore 5 del mattino, la 5a Commissione del Senato aveva dato mandato al relatore di riferire in Aula sulla conversione in legge del il quale è stato ampiamente modificato rispetto al testo iniziale. Tra poco, quindi, si voterà si voterà la fiducia annunciata da giorni. Il testo del disegno di legge è stato depositato ieri sera, ma sentivo che ancora la 5a Commissione ha dovuto rimetterci mano per degli errori. Questa situazione costringe a votare una fiducia sulla fiducia, al buio, e si ripresenta puntualmente, perché è conseguenza della incostituzionale torsione della funzione della decretazione d'urgenza che, secondo la Costituzione, signor Presidente (e la ringrazio per l'ascolto), dovrebbe avere oggetto, se non unitario, almeno omogeneo. Così come, rispetto al decreto-legge, dovrebbe essere omogenea la legge di conversione. Per queste ragioni, a settembre, il Presidente della Repubblica, promulgando il il decreto semplificazioni, ha avvertito l'esigenza di ribadire che, nel corso dell'esame delle leggi di conversione, non possono essere inserite «norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza». Infatti questa prassi priva il singolo parlamentare, attraverso il meccanismo della fiducia, della reale possibilità di esaminare i provvedimenti e i suoi effetti nell'ordinamento, e quindi della possibilità di migliorare il provvedimento. In queste condizioni il Parlamento non può seriamente esprimere un voto in scienza e coscienza. Già la Corte costituzionale, con riferimento all'approvazione del bilancio 2018, che fu portato all'approvazione del Senato, e della Camera poi, con una procedura che evidenzia una certa continuità procedurale tra i due Governi Conte, ebbe a stigmatizzare che quelle modalità procedimentali possono in concreto elidere in modo rilevante le prerogative costituzionali del singolo parlamentare rispetto alla funzione di rappresentanza che egli ha della Nazione che gli è attribuita e che, senza il presupposto della responsabilità e della conoscenza, non trova corretta espressione. La recidivante violazione costituzionale oggi ci impone, nonostante la bontà di alcune misure contenute nel provvedimento, di astenerci dal voto per senso di responsabilità verso parte degli italiani che necessitano di quelle provvidenze: per non danneggiarli quindi. Senza aver potuto valutare il merito del testo approfonditamente e con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

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 104.

L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2,

Signor Presidente, onorevoli senatori, considero sempre importante il momento di confronto parlamentare, così come disposto dal decreto-legge E lo considero tale in modo particolare in questo passaggio della crisi epidemiologica che stiamo vivendo, che vede un'evoluzione costante, e penso che il confronto in Parlamento sull'analisi dei dati visione della situazione non possa che far bene, arricchire la nostra democrazia e anche aiutarci rispetto alle misure che dobbiamo mettere in campo.

del Ministero della salute, delle Regioni e dell'Istituto superiore di sanità. Il quadro credo sia sotto gli occhi di tutti: quello globale è ancora molto complesso (abbiamo superato i 35 milioni di casi confermati e certificati sul piano mondiale); come è noto, negli ultimi giorni è stato superato il numero di un milione di vite spezzate e, quindi, un milione di persone ha perso la vita. Questo è il dato mondiale con cui abbiamo a che fare. Il Centro europeo per la sorveglianza e il controllo delle malattie ogni settimana ci offre invece un'analisi precisa e puntuale sull'evoluzione epidemiologica in ogni singolo Paese dell'Unione.

ci dà alcuni numeri che credo siano utili per istruire la discussione che oggi va fatta in Parlamento: Spagna, 319 casi su 100.000 abitanti Francia, 246; Olanda, 243; Belgio, 220; Gran Bretagna, 163.

in Europa, ma che, se confrontati in una dinamica evolutiva delle ultime settimane, segnalano come in tutti questi Paesi europei ci sia una tendenza molto significativa alla crescita e al peggioramento dei dati epidemiologici. Il nostro Paese, con il numero 45, è ancora molto al di sotto della grande maggioranza di quelli europei, ma la tendenza è in crescita e ci richiede grandissima attenzione. La mia opinione - e questo è il punto di partenza del ragionamento che voglio offrire all'Assemblea del Senato - è che siamo ad un cambio di fase nell'evoluzione epidemiologica europea e del nostro Paese. E quando parlo di un cambio di fase, intendo che in tutti i Paesi che ho provato velocemente a citare, fino a un certo punto, cioè fino alla fase precedente, abbiamo avuto una tendenza ad allargare le misure e a lavorare per un rientro alla normalità, con questo cambio di fase si torna a intervenire con misure che hanno una connotazione di natura restrittiva. Il peggioramento è in corso in tutti i Paesi europei, nessuno escluso, anche se i numeri - come avete visto - sono diversi. I numeri ci dicono oggettivamente che l'Italia in questo momento, insieme alla Germania, è il grande Paese europeo che ha i dati migliori. Ma, attenzione, guai ad illudersi e guai a pensare che, sulla base di questi dati, noi siamo fuori da rischi o fuori da pericoli.

mentre la Gran Bretagna (un altro grande Paese europeo) ha 12.500 casi solo nella giornata di ieri e mentre in alcune grandi e importantissime città europee (penso alla città di Parigi) nella giornata di ieri

alla città di Madrid) già da diversi giorni c'è una forma cauta di *lockdown*, e a oltre un milione di persone viene detto che non si può uscire di casa se non per andare a scuola o al lavoro, non dobbiamo immaginare che, di fronte a una descrizione del clima e della situazione europea di questa natura, noi possiamo sentirci fuori pericolo. I dati italiani segnalano la stessa tendenza, anche se con numeri ridotti rispetto a quelli che vediamo negli altri Paesi. La tendenza è netta, chiara e non equivocabile: sono nove settimane consecutive che i nostri numeri crescono. E con la realtà, come sempre, bisogna fare i conti.

abbiamo avuto una sostanziale concentrazione dell'epidemia in un ambito territoriale molto raccolto e molto chiaramente identificato. identificato. Nei mesi difficili di marzo e aprile, e poi anche nella fase immediatamente successiva, l'epidemia è stata concentrata territorialmente in un pezzo di Paese, in modo particolare la Lombardia e alcune importantissime Province del Nord Italia. Nel resto del Paese la capacità penetrante del virus è stata oggettivamente molto limitata e i numeri dell'analisi sierologica che abbiamo svolto grazie al lavoro prezioso dell'Istat e della Croce Rossa ci hanno consegnato questa fotografia.

Ora c'è una grande novità: la crescita è generalizzata in tutti i territori del nostro Paese. In questo momento non c'è il problema su un territorio, mentre il resto del Paese può sentirsi in qualche modo fuori pericolo. I numeri sono più contenuti, ma crescono in maniera significativa in ogni angolo del nostro Paese. E questo richiede grandissima cautela, grandissima attenzione e un impegno particolare da parte di tutte le istituzioni. La mia opinione è che, sulla base di queste valutazioni, servirà ancor di più quel raccordo costante, continuo e - io credo - proficuo che c'è stato nei mesi precedenti tra le Regioni e lo Stato. Anche ieri sera c'è stata una riunione con tutte le rappresentanze delle Regioni italiane e ve ne sarà un'altra nelle prossime ore, subito dopo la chiusura di questo confronto parlamentare, per condividere le misure importanti che abbiamo di fronte a noi. Le Regioni potranno prevedere misure più restrittive - alcune lo stanno già facendo - ma è particolarmente decisivo in questo momento avere un livello molto significativo di coordinamento tra pezzi delle istituzioni repubblicane. In buona sostanza, sulla base di queste prime valutazioni, voglio affermare che l'Italia oggi ha un vantaggio rispetto agli altri Paesi: i sacrifici fatti, i comportamenti delle persone, le misure dure attuate nella nostra comunità nazionale hanno consentito oggi all'Italia di avere numeri più bassi rispetto a quelli di tanti altri Paesi europei, ma non siamo fuori pericolo.

prima di tutto del nostro Servizio sanitario nazionale, delle donne e gli uomini del nostro Servizio sanitario nazionale, che non smetteremo mai di ringraziare per il lavoro straordinario che hanno fatto e che continuano a svolgere ogni giorno.

e cioè che i risultati - compreso qualche risultato positivo che ho provato a enucleare nella differenza rispetto ad altre realtà europee - non sono mai acquisiti per sempre. Dobbiamo essere nettissimi e dirci la verità su questo punto: i risultati si conquistano ogni giorno e ogni giorno vengono rimessi in discussione. È per questo che credo che la linea che debba guidarci nelle prossime ore e settimane debba essere, ancora una volta, la linea della prudenza, quella linea che finora ci ha guidato a questi effetti e agli attuali risultati. Per questa ragione di fondo, per questa ragione fondamentale, penso sia giusta la scelta del Governo - già resa pubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri - di voler prorogare lo stato d'emergenza al 31 gennaio Ritengo questo atto pienamente corrispondente alla fase epidemiologica che stiamo attraversando. L'impalcatura istituzionale connessa allo stato d'emergenza ci ha consentito di gestire la fase che abbiamo finora attraversato, ed essa è costruita attorno alla centralità della Protezione civile, ai suoi poteri di ordinanza, al ruolo del commissario straordinario e naturalmente al ruolo fondamentale del Comitato tecnico scientifico, che ci ha accompagnato puntualmente nelle scelte che abbiamo compiuto a livello di Governo, a livello di Regioni e anche nell'ausilio ai soggetti sociali rispetto alle misure nella fase di convivenza in cui ancora siamo. La mia opinione è che, pur tra mille difficoltà, pur dentro una complessità che nessuno pensa mai di non considerare adeguatamente, l'impalcatura istituzionale che ci siamo dati sin dai primi giorni della crisi sanitaria è un modello che ha funzionato e che ci ha consentito una maggiore rapidità di intervento dinanzi alle necessità che si sono presentate. Permettetemi anche in questa sede di ricordare che, dal 2004, nel nostro Paese, ci sono state ben 154 dichiarazioni dello stato d'emergenza, e in ben 84 occasioni lo stato d'emergenza è stato prorogato. Se mi è consentita un'ulteriore riflessione, vorrei segnalare come di solito, nella storia del nostro Paese, lo stato d'emergenza si costruisce su eventi che hanno una determinazione temporale molto puntuale. Di solito lo stato d'emergenza viene dichiarato per un terremoto, per un'alluvione, cioè per eventi che sul piano temporale iniziano e finiscono in un ambito puntualmente delimitato. caso siamo oggettivamente di fronte ad un fatto nuovo, inedito nella storia del nostro Paese: non un evento che inizia e finisce in un arco temporale breve e delimitato, ma un evento dinamico, che è iniziato in un determinato momento e che evidentemente non si chiude con una facilità e con una limitatezza, che può essere paragonabile ad altri tipi di eventi. Per queste ragioni io ritengo che sia appropriata adeguata la scelta che stiamo per compiere di allungare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Voglio venire

Consiglio dei ministri, l'orientamento del Governo è di continuare a puntare sulle tre misure fondamentali, che abbiamo ormai fatto diventare le tre regole guida, della iniziativa di contrasto al Covid-19. Le tre regole fondamentali sono quelle che noi abbiamo appreso in questi mesi come regole auree per provare a contrastare il Covid-19. La prima è l'utilizzo delle mascherine. L'utilizzo delle mascherine è la prima regola essenziale; tutta la comunità scientifica mondiale ritiene che questo sia lo strumento principale con il quale provare a contrastare la diffusione del virus. L'orientamento del Governo è quello di estenderne l'utilizzo, rafforzando chiaramente anche questo messaggio al Paese, anche nei luoghi e negli spazi aperti, a prescindere dai limiti orari, che invece finora sono stati vigenti. Noi riteniamo che questa sia una misura consona, appropriata, che può aiutarci a contrastare il virus e che dà anche un messaggio positivo al Paese rispetto al necessario innalzamento della soglia di attenzione in questa nuova fase che ho provato ad indicare. In modo particolare, permettetemi di dirlo, diventa particolarmente decisivo insistere sull'utilizzo delle mascherine in tutte le occasioni in cui si incontrano persone non conviventi. I dati che stiamo riscontrando nelle ultime settimane segnalano che il più alto livello di diffusione del contagio è tra le relazioni più strette, le relazioni personali, le relazioni amicali, le relazioni familiari. Quindi il messaggio deve essere molto chiaro e molto netto: in ogni occasione in cui si può incrociare una persona non convivente sotto lo stesso tetto è fondamentale l'uso della mascherina, che è la prima arma che abbiamo per contrastare il virus. La seconda regola fondamentale, come sapete benissimo, è quella che riguarda il distanziamento di almeno un metro e il divieto di assembramenti. Anche questa è una regola che dobbiamo provare a far rispettare il più possibile. La norma è già vigente, quindi non c'è bisogno di un intervento normativo ulteriore su questo ambito, ma credo che invece ci sia bisogno - ed è intenzione del Governo produrre uno sforzo su questo terreno - di innalzare il livello di attenzione. le norme sugli assembramenti esistono, ma dobbiamo aumentare il livello dei controlli affinché le norme vigenti vengano compiutamente e pienamente rispettate. Il terzo punto di queste regole essenziali ha a che fare con il rispetto delle norme igieniche fondamentali e, in modo particolare, con il lavaggio delle mani.

Non c'entra nulla la politica, non c'entra nulla la destra, non c'entra nulla la sinistra: sono regole essenziali che la comunità scientifica mondiale ci offre e io credo che dovremmo tutti seguirle senza alcuna distinzione. Non avrebbe senso distinguersi su una indicazione di natura scientifica, che oggi risulta essere l'arma più forte per provare a reggere contro il contagio. Rispettare queste regole è davvero essenziale perché ci può consentire di gestire questa fase di transizione. Gestirla significa soprattutto, dal mio punto di vista, creare soprattutto le condizioni perché le strutture del Servizio sanitario nazionale non possano risentire di una pressione troppo pesante, quanto i numeri del contagio hanno evidentemente, poi, una ripercussione sui nostri ospedali e sul lavoro del nostro personale sanitario ed è lì che si può innescare una dinamica che può poi diventare difficile da controllare. Anche in questo caso si tratta di numeri, perché i numeri contano e devono aiutarci nel lavoro che dobbiamo compiere. Oggi in Italia ci sono 58.900 persone risultate positive al test.

Abbiamo 3.487 persone ricoverate nelle nostre strutture ospedaliere con sintomi e 323 posti letto in terapia intensiva occupati a causa del Covid.

Vi ho detto in più occasioni che abbiamo stanziato più risorse sul Servizio sanitario nazionale negli ultimi cinque mesi che negli ultimi cinque anni. Sulle terapie intensive, ad esempio, il cosiddetto decreto rilancio, che le Camere hanno convertito, ha disposto un investimento tale da aumentare del 115 per cento i posti letto. Si tratta di un lavoro che stiamo facendo in piena sintonia con le Regioni. Fornisco però questi numeri perché dobbiamo avere chiara la tendenza: nel momento più difficile, ci sono stati oltre 4.000 posti letto impegnati da persone a causa del Covid. Oggi, che siamo a 323, è chiaro che siamo messi molto meglio rispetto ai mesi più difficili, ma non dobbiamo assolutamente far finta di non vedere che c'è un'altra verità, in quanto durante i mesi d'estate eravamo a 30 posti occupati in terapia intensiva, mentre oggi siamo a 323. Questo significa che abbiamo una situazione che in questo momento è sostenibile, ma c'è una tendenza che va analizzata con la massima attenzione, la quale ci richiede un atteggiamento di grande prudenza e maturità. Tra l'altro, una novità importante di questa diversa stagione del Covid, di questa fase di seconda ondata dentro cui tutta l'Europa evidentemente è l'età delle persone contagiate. Uno degli elementi del minore impatto del Covid sulle strutture sanitarie ha che fare con l'età mediana delle persone che sono contagiate. In questo momento in Italia l'età mediana è di quarantuno

È chiaro che questo è un punto di differenza fondamentale perché il Covid non ha lo stesso effetto, in termini di ricaduta e di peso sulla pressione sanitaria, sulle persone di età più giovane rispetto a chi, invece, ha qualche anno in più. anche da questo punto di vista vi segnalo una tendenza: nel mese di agosto l'età mediana era arrivata a trentuno anni, Quindi, anche sul piano dell'età mediana anagrafica, la tendenza delle ultime settimane è di una crescita comunque significativa che va osservata con grande attenzione. Non vi è dubbio che in queste ore - soprattutto da qui ai prossimi mesi autunnali e invernali, che sono non facili (mi ci soffermerò alla fine) - abbiamo bisogno di tenere l'attenzione più alta possibile soprattutto sui soggetti fragili, ma è evidente che dentro le relazioni intrafamiliari è molto facile che anche dalle generazioni più giovani il *virus* possa trasferirsi a quelle meno giovani. Ancora, in queste ore stiamo ponendo la massima attenzione possibile sulle scuole e sulla sfida che il Paese sta affrontando della riapertura delle scuole. in più occasioni un tema credo condiviso tra maggioranza e opposizione è stato quello della necessità di un'attenzione particolare sulle questioni della scuola e di una loro riapertura in sicurezza. Penso che sia stata una scelta importante e giustissima quella di far ripartire le scuole, è evidente che abbiamo bisogno di un monitoraggio che sia il più accorto possibile. È chiaro che non abbiamo trascorso un tempo sufficiente per esprimere un giudizio definitivo e compiuto. Com'è noto le scuole, in una parte maggioritaria del Paese, hanno riaperto il 14 settembre, ma in un'altra parte significativa hanno riaperto soltanto nell'ultima decade di settembre. I primi dati che ricaviamo e le prime analisi che ci arrivano in modo particolare dall'Istituto superiore di sanità mostrano una sostanziale tenuta del mondo della scuola. Non è la scuola in questo momento il luogo più problematico sul piano del trasferimento e della diffusione del contagio. di esprimere un sentimento di gratitudine per il lavoro straordinario, in un clima difficilissimo e inedito per tutti, che è stato fatto in modo particolare dagli insegnanti, dai presidi, dal personale scolastico e anche dalle famiglie e dai genitori che si trovano si trovano a dover affrontare problemi inediti, senza precedenti. *(Applausi)*. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno pensa di avere la perfezione in mano. È chiaro che siamo di fronte alla gestione di un problema nuovo ed enorme, ma posso dire che che in queste primissime settimane i segnali sono incoraggianti e mostrano una tenuta del mondo della scuola su cui dobbiamo continuare ad investire il più possibile. Lo ribadisco solo un istante: la mia personale opinione è che la sfida più strategica è e sarà sempre quella di una relazione organica, compiuta, strutturata e non episodica tra il Servizio sanitario nazionale e il sistema scolastico: una relazione che è esistita nella storia del nostro Paese,

per rafforzare la nostra capacità di *testing*, perché è un'arma decisiva nella fase che stiamo attraversando. L'ultima volta che sono stato in quest'Aula avevo annunciato che eravamo riusciti a superare la soglia dei 100.000 tamponi al giorno. Era circa un mese fa oggi posso dire (è un dato che ormai conoscete tutti) che abbiamo superato nella passata settimana la soglia dei 120.000 tamponi al giorno. Sono numeri importanti che segnalano uno sforzo che stiamo mettendo in piedi, ma dobbiamo ancora insistere, perché la la capacità di *testing* e di tracciamento è un'arma importante che il Paese ha in questa fase di transizione difficile. Abbiamo, tra l'altro, iniziato ad usare com'è noto - non solo i test classici, quelli del *gold standard* per la diagnosi che sono i test molecolari sull'RNA, ma abbiamo iniziato ad usare, con la mia ordinanza del 13 agosto negli aeroporti e con l'ultima circolare del Ministero della salute anche fuori dagli aeroporti, dove c'è particolare necessità di essere rapidi (penso esattamente alle scuole e ai luoghi della formazione), anche i test antigenici. L'esperienza negli aeroporti è stata positiva e ci ha dato segnali incoraggianti sull'affidabilità di questo tipo di test e quindi l'opinione del Governo, soprattutto dei nostri scienziati, è che possiamo farne un utilizzo più diffuso. Questo è importante, perché la rapidità di risposta è un grande tema che dobbiamo necessariamente affrontare. La scienza evolve e oggi ci dà strumenti che qualche mese fa non avevamo. Il nostro auspicio è che tra qualche settimana ci dia strumenti ancora più evoluti, ancora più fini fini e più capaci di rispondere alle nostre esigenze. Per esempio, sul piano del *testing* il mio auspicio è che si possa, in un tempo congruo chiaramente e nel rispetto di tutte le procedure formali vigenti, arrivare anche ad un utilizzo dei test salivari significativo. I test salivari possono essere importanti perché è evidente che hanno una modalità esecutiva meno invasiva, a differenza del tampone che ha comunque una modalità abbastanza invasiva. Il test salivare da questo punto di vista può essere particolarmente utile, in modo particolare per le fasce anagrafiche relative ai più piccoli. Io sono convinto - lo ribadisco ancora in quest'Aula che la scienza ci darà risultati importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. C'è un lavoro senza precedenti della comunità scientifica internazionale a tutti i livelli.

Il vaccino in questione è il cosiddetto vaccino di Oxford, prodotto da AstraZeneca, su cui l'Italia ha costruito tra l'altro la prima intesa con Francia, Germania e Olanda nel mese di giugno, e su cui, come noto, c'è anche un impegno importante di alcune realtà del nostro Paese. In modo particolare, rispetto a questo vaccino, il vettore virale viene fatto dall'IRBM di Pomezia e l'infialamento viene fatto dalla Catalent di Anagni. Io credo che sia un fatto importante che dentro questa sfida internazionale, il nostro Paese sia in prima linea perché il vaccino possa essere al più presto un bene pubblico di tutti, capace di dare la risposta che tutta la comunità internazionale aspetta. Se ne parla meno, ma passi in avanti importanti si stanno facendo anche sul terreno delle cure; in modo particolare le cure che sembrano avere risultati più incoraggianti sono quelle connesse agli anticorpi monoclonali. Anche da questo punto di vista c'è un lavoro prezioso che viene portato avanti da numerosi scienziati italiani e che ci auguriamo possa essere valorizzato. Nel decreto di agosto,

C'è infatti una posta di bilancio di 80 milioni di euro per il 2020 e di 300 milioni di euro per il 2021, esattamente su questo settore di ricerca che è essenziale e su cui il nostro Paese deve necessariamente continuare ad essere all'avanguardia. Come è noto, io ho molta fiducia. Io penso che la comunità scientifica mondiale ci darà in un tempo congruo strumenti e armi per poter vincere questa sfida. L'umanità, il mondo, l'Europa e l'Italia vinceranno la sfida del Covid. La verità però è che abbiamo bisogno ancora di tempo; dinanzi a noi ci sono mesi non facili perché questi strumenti non arriveranno domani mattina, saranno, nella migliore delle ipotesi, nella nostra disponibilità nel giro di alcuni mesi. Si tratta di un tempo significativo, non è un tempo breve e, allora, il punto di fondo che voglio sottoporre all'attenzione di quest'Aula è la capacità di resistenza che noi dobbiamo avere.

vede, ma ha bisogno ancora di un lavoro di alcuni mesi, in cui le uniche armi che abbiamo davvero per combattere continuano ad essere il comportamento delle persone, le misure del Governo nazionale e dei governi regionali, e il tracciamento, che è molto importante. Permettetemi anche in quest'Aula di esprimere gratitudine per gli editori e i media del nostro Paese che hanno dato una spinta all'*app* Immuni che negli ultimi giorni sta avendo un risultato positivo in termini di *download*. Naturalmente dobbiamo poter puntare sempre di più sul nostro Servizio sanitario nazionale. In questi mesi è l'arma più importante che abbiamo; le nostre donne, i nostri uomini, le persone che lavorano ogni giorno pancia a terra per affrontare e combattere il virus. Sono stato pochi giorni fa nella Commissione igiene e sanità del Senato ed ero stato, pochi giorni prima ancora nella Commissione affari sociali della Camera, per provare a offrire anche un disegno di potenziale riforma e rilancio del Servizio sanitario nazionale. Penso che ciò sia particolarmente importante e mi auguro si sviluppi a un certo punto una discussione in Aula, oltre che nelle Commissioni, sul tema di come immaginiamo il Servizio sanitario del futuro. È l'arma più importante che abbiamo, è la pietra più preziosa del nostro sistema Paese. E ora arriva una straordinaria opportunità: è la lezione del Covid-19, cioè provare a riformarlo, a cambiarlo, a rafforzarlo, non in una fase restrittiva, ma in una fase in cui ci sono più risorse. Io credo che questa sia una grandissima possibilità, che dobbiamo assolutamente raccogliere, a partire dalle nuove linee dei finanziamenti europei.

ad uno snodo e che bisogna necessariamente alzare il livello di guardia. Questo è il messaggio fondamentale che noi vogliamo provare a dare con i provvedimenti che metteremo in atto nelle prossime ore. Dobbiamo alzare il livello di guardia. primo punto è che la sicurezza sanitaria è la premessa di ogni ripartenza economica. Io insisterò con tutte le energie che ho su questo punto. È sbagliatissimo cedere a un'impostazione culturale che fa pensare a tanti che avere meno lacci, meno vincoli sanitari, possa aiutare il Paese a correre di più. La mia opinione è che non ci sia nulla di più sbagliato ed è esattamente all'opposto. Se vogliamo mettere nelle condizioni il Paese di ripartire davvero, la premessa è vincere la battaglia sanitaria.

io credo, come vi ho detto con grande onestà e con grande trasparenza, che i prossimi mesi non saranno facili, per le ragioni che ho descritto. In un contesto mondiale europeo molto complicato, non possiamo farci illusioni. Non possiamo pensare che sarà una passeggiata. In questa sfida dei prossimi mesi, in attesa del vaccino e in attesa delle cure, noi abbiamo bisogno che il Paese ritiri fuori il meglio di sé. Voglio dire fino in fondo quello che penso. Io penso che, nei mesi più difficili, L'Italia - non il Governo, ma l'Italia - abbia dimostrato di essere un grandissimo Paese. Le sue donne, i suoi uomini, la Protezione civile, le Regioni, le istituzioni a tutti i livelli, i Comuni e poi ancora le reti di volontariato e di solidarietà: abbiamo dimostrato di essere un grande Paese, che in queste ore viene visto con attenzione anche da altri Paesi in giro per il mondo. il mondo. Dobbiamo recuperare quello spirito. Io penso che, nei mesi che mancano da qui a quando davvero vedremo la luce, noi abbiamo bisogno di recuperare lo spirito che ci ha accompagnato a marzo, ad aprile, a maggio. Quel grande spirito di unità, con un Paese che ha avuto la forza di stringersi a coorte e di vincere la sfida drammatica che in quei momenti stava arrivando. Io penso che nei prossimi mesi dovremo esattamente recuperare quello spirito e unire l'Italia. Nessuno deve rimanere fuori. C'è bisogno di unire l'Italia, per dimostrare, ancora una volta, che l'Italia è davvero un grande Paese.

Ha evocato una serie di suggestioni su cui non possiamo che convenire, con un profondo - ahimè - profondissimo limite, che anche la sua garbata eloquenza non è riuscita a colmare.

apro e chiudo un inciso. Signor Ministro, lei ha ricordato stati di emergenza settoriali, non stati di emergenza generali. Qui parliamo di uno stato di emergenza che, non tanto tempo fa,

Mi creda, signor Ministro, lei ha di fronte delle persone collaborative, lo abbiamo dimostrato anche se - lo ripeto ancora una volta - risultano quasi urticanti queste continue evocazioni di collaborazione e richiesta di solidarietà da parte di un Governo che, a parte qualche piacevolissimo caffè a Palazzo Chigi, non ci ha particolarmente coinvolti nella sua attività di gestione dell'emergenza *(Applausi)*, nonostante noi avessimo e abbiamo ancora utilissime ricette sanitarie, economiche e di economia della conoscenza - probabilmente il tema più importante di questi tempi - per far ripartire velocemente il Paese. Signor Ministro, io ritengo davvero che non sia possibile che lo stato di emergenza significhi inserire dei contenuti così importanti per tutti noi. Ciò di cui stiamo parlando, lo ripeto, lo dice la lo dice la Nota di aggiornamento al DEF in quella parte relativa agli scenari possibili della pandemia, in cui si dice che saranno possibili altre chiusure selettive

ma non così, non in questo modo, non illudendo gli italiani, signor Ministro, che lo stato di emergenza significhi maggiore sicurezza. al Governo dovreste dimostrare, come tutti gli altri Governi di Europa, di essere in grado di governare questo Paese con gli strumenti ordinari, non con le leggi speciali e con gli editti che tagliano fuori l'unico organismo che sia legittimato a tagliare i diritti di libertà, cioè il Parlamento.

che un atto unilaterale del Governo faccia aggio su un organo come il Parlamento che rappresenta tutti gli italiani e quando si prendono provvedimenti che riguardano tutti gli italiani c'è un'unica casa in cui questi provvedimenti devono essere discussi: questa. *(Applausi)*. Lo dico non solamente a lei, signor Ministro, ma anche ai colleghi della maggioranza, che non devono consentire, per problemi di gestione delle dinamiche governative, che questi diritti siano sottratti a questo organismo, a questo organo, a questo collegio per sempre. La prego, signor Ministro, lei è persona competente, trasferisca a chi di dovere questo pensiero. Non è possibile, per portare a casa un risultato oggi, privare il Paese della doverosa separazione dei poteri domani e per sempre. *(Applausi)*. Anche questo è il futuro del Paese. Lei ha detto di voler ringraziare gli operatori sanitari e gli operatori della scuola. Lo deve fare veramente, perché soprattutto per gli operatori della scuola, signor Ministro, non è andato tutto bene. Dobbiamo ringraziare tutti eccetto il ministro Azzolina, e non è poca cosa, signor Ministro. Abbiamo avuto sei mesi per predisporre dei protocolli di sicurezza. Lei ha ragione quando dice che si sta facendo il possibile, ma il possibile, quando si richiedono leggi speciali e pieni poteri, non è sufficiente. Lei sa bene che esistono dei problemi legati a presidi sanitari che nella scuola non sono mai stati predisposti. Lei sa che esistono problemi legati alla gestione di problemi sanitari che da adesso in poi diventeranno sempre più gravi, perché come ci avete detto tante volte da qui ad aprile cinque milioni di persone, signor Ministro, signor vice Ministro, si ammaleranno di malattie virali respiratorie che non sono Covid, ma che potranno sovrapporsi al Covid, di cui i medici non saranno in grado di fare diagnosi e dove andranno questi malati? malati? In ambulatori pubblici, privati, pronto soccorso, dai medici di base? Avete organizzato dei protocolli di sicurezza per tutto questo? Noi ve lo stiamo chiedendo da sei mesi. Vi stiamo chiedendo da sei mesi di organizzare il sistema scuola, quantomeno predisponendo delle sicurezze anche anche strutturali. È servito a qualcosa cambiare i banchi? Avete visto delle scene terribili: banchi a rotelle che cozzavano gli uni contro gli altri, alla faccia del distanziamento sociale. Vediamo assembramenti fuori dalle scuole. Signor Ministro, non possiamo dire che quando va tutto bene è merito del Governo e quando non va tutto bene, come adesso, è colpa degli italiani. *(Applausi).* Lei solo ha riconosciuto che non è così, ma il suo Presidente del Consiglio e il suo Governo no. Siamo intellettualmente onesti. Signor Ministro, ancora una cosa. Noi ci rifiutiamo - e combatteremo fino all'ultimo respiro - di consentire che lo stato di emergenza venga esteso a tutti gli italiani e alle loro libertà fondamentali, e che ci sia un ordinario prelievo fiscale, a partire dal 15 ottobre, con 9 milioni di cartelle che partiranno ai danni di contribuenti che non stanno guadagnando o stanno guadagnando molto meno. Noi chiederemo e continueremo a chiedere la proroga di tutte le scadenze fiscali, dei pignoramenti degli stipendi e delle pensioni fino al 31 gennaio 2021. Questo è doveroso. Uno Stato che chiede soldi a chi non guadagna o a chi guadagna meno non per sua colpa è uno Stato tiranno *(Applausi),* e noi non vogliamo essere complici di uno Stato tiranno. Signor Ministro, noi abbiamo molte cose da dire e le diremo nei nostri interventi. Lei ha capito che lo stato di emergenza non ci piace per un motivo specifico. Ci sta raccontando oggi delle cose con una finzione che non ci è mai piaciuta, perché lei ci viene a raccontare qualcosa su cui noi diciamo altre cose di cui lei non terrà conto. conto. Il Governo farà comunque il suo atto unilaterale, indipendentemente da quello che le diremo noi nelle due ore successive. *(Applausi).* Questa è una presa in giro, signor Ministro, prima di tutto del Governo, ancor più che del Parlamento. Vi prendete in giro da soli. Noi chiediamo e pretendiamo che quello che state facendo, lo facciate con l'unico strumento previsto dalla Costituzione per la necessità e l'urgenza: i decreti-legge. Colleghi, signor Ministro, la Costituzione non è un orpello che si mette da parte quando non si ha convenienza ad usarla. La Costituzione è sempre e per sempre, e la Costituzione ha predisposto chiari strumenti per l'emergenza. Non chiedeteci più di collaborare facendo gli osservatori non partecipanti. Ve lo abbiamo detto tante volte e ve lo ripetiamo: noi ci siamo per collaborare, per lavorare insieme, ma per noi la collaborazione non sarà mai obbedienza. *(Applausi).*

la Lega ha sempre sostenuto che per contrastare la pandemia, al di là della questione stato di emergenza sì-stato di emergenza no, quello che davvero conta, la vera sostanza, è sapere se il Governo è pronto ad affrontare questa situazione, sì o no. Si è preparato il Governo? Noi l'abbiamo chiesto con un'interrogazione il 7 luglio: era abbastanza scontato che ci poteva essere o che ci saremmo potuti trovare di fronte ad una seconda ondata, ad una recrudescenza del virus. Quindi dobbiamo capire se il Governo è pronto. Sullo stato di emergenza, mi perdoni, signor Ministro, senza entrare in polemica. I colleghi del centrodestra l'hanno abbondantemente messo in evidenza, però ultimamente uno spunto di riflessione non solo per lei e per il Governo, ma per tutto il Parlamento, è venuto dall'intervento che ha fatto il costituzionalista Sabino Cassese, il quale ha detto che «l'emergenza non c'è,

la vita è ricominciata, il virus circola, si sapeva che ci sarebbe stato questo. Lo stato d'emergenza «serve soltanto perché all'interno della macchina statale c'è un'impotenza nell'affrontare i problemi ordinari». Sostanzialmente, serve per sveltire quelle procedure - dice Sabino Cassese - che non si ha la capacità di sveltire in modo ordinario.

almeno le persone cosiddette a rischio, le persone più fragili e più deboli avranno la possibilità di vaccinarsi? Queste sono

c'è un rallentamento sulle altre patologie. Ci sono 1,4 milioni di *screening* in meno; addirittura ci è stato detto che, con diagnosi tardive, il rischio è che aumenti la mortalità dei pazienti. Questo è avvenuto nei primi cinque mesi del 2020.

altre patologie. Stiamo lavorando per garantire che non ci siano liste d'attesa infinite e che gli *screening* si svolgano? Stiamo lavorando affinché gli ospedali possano riprendere un ordinario lavoro anche su tutte le altre patologie? Altra questione

sicuramente a partire da fine ottobre o inizi di novembre, siamo sicuri che i genitori non correranno tutti al pronto soccorso per chiedere di fare immediatamente il tampone e verificare se si tratti o meno Covid-19? Il sistema di medicina territoriale di cui si è tanto parlato è stato potenziato? I medici di base sono pronti ad affrontare la situazione, ad andare a visitare i bambini direttamente nelle case, presso le famiglie? Abbiamo sviluppato questo tipo di modalità? Abbiamo fatto scorte

dare una visione dei dati più trasparente, come avevamo già chiesto nell'ultima discussione. Signor Ministro, cerchiamo di capirci: ci sono giornali che hanno titolato, «dati mai così alti», «come nel mese di aprile», ricordando il periodo del *lockdown*.

che non ci sia un dato scientifico che ci dica, sulla base dei tamponi eseguiti, quanti sono esattamente gli asintomatici? *(Applausi)*. Non conosco questo dato, ma gli italiani hanno il diritto di conoscerlo!

Questo è il ragionamento che volevo fare. è giusto essere prudenti, ma anche avere buon senso. Infatti, se continuiamo con questi messaggi che terrorizzano la popolazione, fra poco, quando cominceranno le prime influenze, la gente per paura starà a casa; non ci sarà un *lockdown* dichiarato, ma di fatto sarà così:

bisogna usare prudenza, mascherine e distanziamento e lavarsi le mani; proteggiamo gli anziani e le persone che hanno particolari patologie, ma diciamo anche che oggi siamo in grado di curare le persone che eventualmente si vogliono ammalare.

Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, a me sembra di avere una strana sensazione di *déjà-vu,* nel senso che molte delle cose che ho sentito dire oggi in questa occasione sono assolutamente analoghe e sovrapponibili a quelle che il Ministro ci ha detto pochi giorni fa e che il Vice Ministro ha riecheggiato nel lavoro della Commissione: sono dati che si ripetono. Potremmo anche dire che *repetita iuvant,* perché tutto sommato sono la descrizione di una situazione e una proposta di interventi. La situazione è quella che è, con indicatori in crescita rispetto al numero dei contagi e dei malati; d'altra parte, le misure

ma tutto questo non può definire, risolvere e in qualche modo concentrare l'intero messaggio che dal Governo arriva attraverso

C'è qualcosa di più che abbiamo bisogno di sapere e mi riferisco perlomeno a tre linee molto concrete di quello che ha detto. In primo luogo, una delle parole chiave che ha utilizzato è «priorità». La salute è una priorità, lo dico io che sono in Commissione sanità da quando sono in Parlamento e sono perfettamente convinta che il tema salute debba rappresentare, nell'economia dello Stato, anche un investimento e non un costo; pertanto, da questo punto di vista, non solo la considero una priorità, ma anche uno di quei famosi diritti tutelati dalla nostra Carta costituzionale con una

Normalmente l'opposizione alza la palla e la maggioranza la schiaccia, nel senso buono del termine: uno alza il livello delle aspettative e l'altro, che rappresenta la maggioranza e quindi dovrebbe avere un senso del realismo più concreto, risponde

svalutando la concretezza dei contenuti che vengono proposti. Pertanto, le ripropongo il tema e le parole chiave "unità" e "collaborazione" ad altri livelli. Per esempio,

come modelli in cui nel territorio le diverse competenze trovano un luogo di dialogo. Ma di questo non abbiamo mai visto nulla nelle proposte operative

"c'è bisogno di questo, stiamo facendo questo e faremo questo". Tuttavia, sappiamo che molto spesso il passaggio attraverso la Conferenza Stato-Regioni riesce a vanificare tutto, perché le priorità percepite a livello regionale di volta in volta sono altre. Mi permetto di sottolineare un'altra cosa importante:

signor Ministro, che ci aspettiamo una risposta ai bisogni di sanità che davvero rifletta quell'unità che invoca, del sapere, della collaborazione e delle forze democratiche, cioè un dialogo operativo e concreto al servizio del paziente, che ci sembra in questo momento manchi un po'.

a marzo eravamo un posto da evitare in tutti i modi, un epicentro da incubo. Oggi siamo un modello di contenimento del virus in grado di dare lezioni al resto del mondo, perché le autorità italiane hanno fatto quello che andava fatto, e rapidamente. Hanno stabilito un *lockdown* durissimo, anteponendo le vite all'economia, attraverso una combinazione di vigilanza ed esperienza medica acquisita dolorosamente, che potrebbe rivelarsi più vantaggiosa anche per l'economia stessa con l'aiuto degli interventi pubblici che hanno sostenuto lavoratori e imprese. Queste, signor Ministro, sono le parole del «New York Times», riferite alla gestione della pandemia in Italia. È così: non eravamo pronti ad affrontare quest'emergenza sanitaria perché il nostro Servizio sanitario nazionale veniva da un decennio di tagli scellerati. Non avevamo posti letto in terapia intensiva, i reparti degli ospedali pubblici erano a corto di personale e le infrastrutture e le tecnologie erano obsolete. In quasi tutte le Regioni mancavano quelle reti di cure primarie e intermedie che servivano a fare da filtro, quindi i medici di medicina generale sono stati i primi a contagiarsi. Hanno dovuto chiudere gli studi, perché non erano attrezzati a gestire una pandemia, non avevano i dispositivi di protezione individuale e non erano stati formati; nelle prime fasi di quest'emergenza abbiamo perso tante vite, spesso perché i pazienti aspettavano a casa per giorni, in attesa di essere sottoposti a tamponi, o venivano curati con terapia sintomatica per poi essere trasportati al pronto soccorso quando insorgeva dispnea, che era segno di un danno polmonare acuto, non sempre reversibile. Troppe le vite perse: 36.000, tra cui molti operatori sanitari, e questi numeri oggi li ripeto perché devono restare impressi nella mente. La storia dev'essere insegnamento per il futuro e non può essere rinnegata. Non è ammissibile che in quest'Aula ancora oggi si parli di complotti, di verità nascoste, di infezione inesistente e di inutilità delle misure di tracciamento e contenimento. Abbiamo sentito parlare di virus clinicamente morto, ma è chiaro che uno che in altri Paesi miete migliaia di vittime non lo è; semplicemente, forse, semplicemente, forse, da noi circolava di meno proprio grazie al *lockdown* messo in atto. Era chiaro che, con la riapertura delle attività, anche i contagi avrebbero ripreso ad aumentare e, di conseguenza, nel tempo sarebbe aumentata la quota di soggetti sintomatici che necessitavano di assistenza medica. Voglio chiarire, rispetto a quanto ha detto il senatore Romeo, che ad aprile facevamo i tamponi a tutti i soggetti sintomatici, quindi è chiaro che la percentuale di positivi era più alta all'epoca. Oggi, invece, il fatto che tra tutte le persone sottoposte a tampone una minima parte sia realmente positiva al virus è indice del funzionamento delle misure di tracciamento che abbiamo messo in atto. Ministro, mi dissocio fermamente da chi strizza l'occhio ai negazionisti per racimolare qualche consenso in più e da chi, per la propria incoscienza, sta mettendo ancora una volta a repentaglio la vita dei miei colleghi medici, degli infermieri e del personale sanitario. Questo Governo e questo Parlamento hanno l'obbligo morale di difendere tutti i cittadini del nostro Paese e mettere in sicurezza la loro salute, che non è un lusso per pochi, ma un bene primario da tutelare. Anche quei cittadini che qualche assessore alla sanità chiama "ordinari" devono poter essere curati nel migliore dei modi e la sanità privata dev'essere una stampella per il servizio sanitario pubblico e non una spugna che drena risorse e scende in campo solo quando ben remunerata. *(Applausi).* I principi del nostro Servizio sanitario nazionale devono essere difesi e tutelati a tutti i costi,

Resteranno per sempre negli occhi di tutti noi le immagini dei senzatetto ammassati nei parcheggi dei centri commerciali negli Stati Uniti o dei poveri in India, arrampicati sugli alberi per sfuggire ai contagi. Anche noi abbiamo barcollato e rischiato di cadere, stremati sotto i colpi della pandemia, ma ne siamo usciti grazie alla resilienza e allo spirito di sacrificio del nostro personale sanitario, mandato a combattere con penuria di mezzi e uomini, su un campo di battaglia reso impervio da politiche scellerate, che per anni hanno perpetrato tagli, trasformando il diritto alla salute in bene per pochi e l'investimento in salute in una spesa sacrificabile. Questo Governo ha fatto sforzi incredibili, chiedendo aiuto - come ha ribadito, signor Ministro - alle menti brillanti dei nostri scienziati, per mettere a punto linee guida e protocolli che guidassero gli operatori sanitari nell'affrontare un nemico che ancora oggi è in gran parte sconosciuto. Ogni giorno i medici, gli ospedali e i funzionari sanitari italiani raccolgono più di 20 indicatori sul virus e inviano questi dati alle autorità regionali che li inoltrano all'Istituto superiore di sanità. Questo modello ci consente di avere una radiografia aggiornata della salute del Paese, su cui poi si basano le decisioni politiche. Partiamo quindi dai dati e da quel metodo scientifico che, in circostanze come questa, è l'unica ancora di salvezza. Prorogare lo stato d'emergenza oggi serve proprio a continuare a rispondere rapidamente in caso di nuovi focolai o di ulteriore aumento dei contagi. Il Presidente del Consiglio ha detto più volte che la salute del popolo italiano viene e verrà sempre prima di tutto e oggi ribadiamo questa scelta di tutela della salute pubblica prima di ogni altra cosa. signor Ministro, bisogna resistere, come ha detto, ma anche guardare al futuro, perché, quando questo finirà, nulla sarà più come prima. Per fare questo, bisogna avere obiettivi definiti e precisi, a breve e a lungo termine. Signor Ministro, a breve termine, per controllare i contagi, serve che la diagnosi sia sempre più tempestiva, per tracciare e isolare tutti i casi positivi. Per fare questo bisogna utilizzare, appena saranno disponibili, i test molecolari rapidi; nell'immediato utilizziamo invece i test antigenici validati, che hanno buona sensibilità e specificità. Serve la presa in carico precoce, domiciliare e territoriale, per monitorare i pazienti attraverso la telemedicina e, se necessario, curarli già alle prime manifestazioni dei sintomi, per evitare complicanze. Per questo è fondamentale che i medici di medicina generale abbiano protocolli e linee guida definiti. Servono ospedali Covid-19, che siano dedicati, perché non possiamo non possiamo più trasformare i nostri nosocomi in focolai né sospendere l'attività ambulatoriale ordinaria. Riprendo quanto detto anche dal senatore Romeo: in questi mesi sono oltre un milione gli esami di *screening* oncologici non effettuati e ciò comporterà un aumento non solo delle diagnosi di cancro, ma anche di mortalità per ritardi nella presa in carico e nella cura dei pazienti oncologici. A medio e lungo termine, invece, signor Ministro, serve un grande progetto di riforma del Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo riorganizzare l'intero sistema di prevenzione pubblica e restituire centralità alla medicina territoriale, spostando l'attenzione dagli ospedali al territorio. ridotta l'ingerenza politica nella gestione regionale della sanità e rafforzato il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo del livello statale. Devono essere ridefiniti i rapporti con la sanità privata: le residenze sanitarie assistenziali devono essere riconvertite in centri di cura e riabilitazione per pazienti che hanno bisogno di cure intensive non praticabili a domicilio, naturalmente sotto la gestione e la vigilanza pubblica. portato avanti senza titubanze il processo di digitalizzazione, attraverso la cartella clinica elettronica e il fascicolo sanitario elettronico. Dev'essere riformato il sistema di emergenza-urgenza territoriale. È giunto quindi il momento di riformare la nostra sanità, per renderla strumento di tutela ed esercizio del diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, mettendo al centro proprio la programmazione, le competenze e la valorizzazione del merito; perché solo con progetti solidi e lungimiranti potremo utilizzare al meglio i fondi del *recovery fund* e quelli reperiti dal *next generation* EU. Non possiamo rischiare di sprecare quest'opportunità e il grande insegnamento che l'imprevedibilità drammatica delle tragedie ci ha riservato. che non basta essere singoli individui, ma bisogna muoversi come squadra, se si è collettività e se ciascuno agisce nell'interesse di tutti. E noi, signor Ministro, siamo certi che lei e questo Governo abbiate a cuore l'interesse dei cittadini italiani e la tutela della loro salute e saremo al suo fianco in questa battaglia, lavorando sempre come squadra in modo costruttivo.

appartenenze politiche competitive tra di noi, perché in questo momento è giusto riconoscere, con obiettività, quando le persone si sono comportate bene nel loro lavoro politico. politico. Ai colleghi dell'opposizione dico che, complessivamente, dovremmo riconoscere che il Governo, nell'affrontare il tema della pandemia da coronavirus, ha lavorato bene. Non dobbiamo avere paura di constatare come, in fondo, i risultati che oggi abbiamo ottenuto siano stati migliori di altri Paesi e non credo che questo debba farci dispiacere. Ciò deve anzi, in qualche modo, renderci orgogliosi, perché è un risultato dell'Italia

che in questo dibattito negazionisti non ne ho sentiti (lo dico anche per essere obiettivi). Credo che in Italia l'opposizione non possa essere identificata con il negazionismo

grazie a Dio, non sono pari a quelli che si registrano a Parigi o Madrid, grazie alle azioni che abbiamo fatto. Qual è il punto che abbiamo di fronte oggi? È cercare di essere fermi e rigorosi, ma equilibrati. Ci sono alcune cose che non riesco a capire e, se le pongo oggi in questo dibattito parlamentare, non è certo per critica, ma perché voglio cercare di dare un contributo come parlamentare. Ad esempio, questa mattina

Lo sport non è un settore che possiamo definire secondario, in quanto è un grande settore che coinvolge l'interesse degli italiani, dà un segno di pseudo-normalità, anche con gli stadi vuoti, e ha grande rilevanza economica. Mi viene

non adottare lo stesso criterio di proporzionalità nelle strutture chiuse, quando poi abbiamo la gente stipata negli autobus o nei treni pendolari (mentre

A Verona possono andare in mille allo stadio, mentre, quando gioca

La stessa cosa vale per gli impianti al chiuso: ho visto che il presidente della mia Regione Bonaccini ha cercato di introdurre criteri che secondo me sono giusti, perché sono improntati alla fermezza: giusti le mascherine, il distanziamento e il divieto di assembramento, ma nello stesso tempo ci vuole ragionevolezza, perché non si può essere omissivi rispetto ai trasporti pubblici e magari duramente repressivi rispetto a eventi sportivi che hanno un grande impatto economico, ma che danno anche il segno di un Paese che, con queste giuste restrizioni che lei ha proposto, torna sulla strada della normalità. Ho dato questo mio contributo augurandomi che

a mio avviso è assolutamente incontestabile l'estensione dello stato di emergenza pandemica al 31 gennaio 2021, come ci propongono il Ministro e il Governo tutto, ma è altrettanto importante che questo tempo venga utilizzato al meglio. Le

e il rafforzamento del sistema sanitario, degli ospedali, dell'assistenza domiciliare e territoriale (come il Ministro ha detto più volte) e della prevenzione in tutte le Regioni, a partire da quelle più deboli. Quindi, servono risorse subito e nei prossimi mesi per mettere a posto la sanità. Invito il Ministro, i colleghi e le colleghe di opposizione e di maggioranza a fare una discussione vera e approfondita sulla necessità di accedere ai finanziamenti del MES sanitario. Sono sicura che le nostre posizioni si avvicinerebbero, a fronte dei vantaggi dell'intera popolazione. Utilizzare al meglio questo tempo significa dare importanza al rispetto per il Regolamento sanitario internazionale, che nel caso delle malattie infettive tiene presente che un virus originato in un Paese può diffondersi ovunque. Il Regolamento dovrà essere aggiornato alla luce del Covid. L'esperienza attuale ci insegnerà cosa fare nel futuro per prepararci a eventuali nuove pandemie. Il Covid-19 potrebbe essere in questo senso un'opportunità che va oltre il disastro creato. Usare bene questo tempo significa mettere a posto la questione dei trasporti, come ricordava bene il presidente Casini. Usare al meglio questo tempo sarà necessario per incrementare i tamponi e il tracciamento.

per effettuarne uno. Dobbiamo usare questo tempo anche per abbattere i tempi d'attesa e per la comunicazione dei risultati, quindi per mettere in sicurezza le persone e le famiglie. Inoltre, dobbiamo essere consapevoli del percorso fatto. All'inizio, i tamponi venivano fatti solo ai sintomatici, mentre gli asintomatici potevano trasmettere il virus. L'abbiamo imparato, per cui aver esteso l'emergenza ha contribuito a capire qual era il vero problema. Molto importante è quello che si sta compiendo nell'ultimo periodo nell'interpretare davvero i risultati più fini e precisi dei tamponi. C'è una certa quantità di italiani che risultano debolmente positivi, perché nel tampone si rivela la traccia dell'RNA e ci si chiede se possano o non possano infettare. È molto interessante che la scienza vada avanti su questo, perché aiuta la politica a prendere decisioni. Il rapporto tra sintomatici

test rapidi, di qualità, di cura e di vaccini. Abbiamo bisogno altresì di rafforzare, aiutare e sostenere la filiera industriale della sanità,

Bisogna istituire una rete nazionale, integrata con quella europea, di centri dedicati allo studio e alla messa a punto di soluzioni terapeutiche, diagnostiche e preventive. Ministro, ci ha assicurato in quest'Aula, nelle comunicazioni del 2 settembre scorso, che ogni passaggio parlamentare mai è rituale e formale, ma è un'occasione utile per raccogliere spunti e suggerimenti dentro una dialettica che possa essere sempre la più proficua possibile, che rende sempre più forte la nostra democrazia. Ha ribadito questo concetto stamattina e, oggi più che mai, il ruolo del Parlamento diventa centrale, se vogliamo agire nella piena consapevolezza e responsabilità non solo della separazione dei poteri, ma anche del loro bilanciamento, soprattutto in stato di emergenza. Noi parlamentari siamo nei territori, raccogliamo e accogliamo le preoccupazioni, le paure e le speranze delle cittadine e dei cittadini,

9 settembre, ho auspicato e sollecitato io stessa la necessità di trovare un terreno comune e uno spazio che consenta la formazione di norme condivise, che evitano a volte una dialettica difficile, distogliendo spesso l'attenzione dalla drammatica portata della gravità del problema, che ha prostrato il mondo intero. Si proroghi quindi lo stato di emergenza nel pieno rispetto dell'equilibrio tra libertà individuale e norme temporanee, non di restrizione, ma di adeguamento razionale, proporzionato ed efficace per per la tutela della salute e di tutte le attività. Chiediamo ai cittadini di rispettare le regole e sul punto, signor Ministro, la seguiamo sempre. Non penso che il Governo, come a volte si dice, tragga per sé o per altri alcun vantaggio dalla decretazione d'urgenza o dalla proroga di uno stato di emergenza fine Chi pensa questo dovrebbe valutare anche il rischio di impopolarità di un Governo che si esporrebbe, se non ve ne fossero realmente e storicamente i presupposti, fondate ragioni e rischi per l'intero sistema Paese. I dati che il Ministro ci ha qui portato e la comparazione con la situazione degli altri Paesi che si trovano, come noi o anche peggio, a gestire l'epidemia, ci impongono serietà, responsabilità e consapevolezza dei nostri ruoli. L'ultimo tema è quello del rapporto tra Stato e Regioni. Ho avuto già altre volte occasione di dire che, a mio avviso, va colmato un vuoto nel nostro ordinamento giuridico, prevedendo una norma che decida in condizioni di epidemia, come ha fatto la Germania. In conclusione, lo stato di emergenza va bene, temperato però dalla rassicurazione che il Governo e il Parlamento insieme devono dare alla popolazione italiana.

purtroppo negli ultimi giorni stiamo assistendo con preoccupazione a una crescita nella curva dei contagi, nei ricoveri ordinari, in quelli in terapia intensiva e anche purtroppo nei decessi, nei numeri dal Ministro stesso. Il Covid-19, nonostante il tentativo di qualcuno di descriverlo come un virus clinicamente morto, è ancora vivo e continua ad avere un impatto drammatico sulle nostre società, sulle relazioni, sulla nostra vita emotiva e sul lavoro. Chiunque in queste ultime settimane abbia lasciato intendere il contrario è irresponsabile e ha diffuso pericolose menzogne. Per comprendere l'entità del problema è sufficiente guardare al di là dei nostri confini, dove la situazione appare fuori controllo. Penso a Parigi e a Madrid, per esempio. Noi abbiamo un atteggiamento di maggiore prudenza e lungimiranza, che ci ha consentito di diventare un modello nella gestione del virus, un modello seppure imperfetto si intende, ma un modello a livello mondiale. Nessuno infatti può negare che gli effetti dell'ondata di ritorno del Covid-19 hanno ad oggi una dimensione diversa rispetto a quella di molti altri Paesi europei. Non sappiamo certamente se ciò che sta accadendo nel resto del continente possa accadere nelle prossime settimane o mesi anche in Italia, ma sappiamo che la nostra capacità di convivere con il virus è un risultato riconosciuto a livello internazionale. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ci ha messo tra i Paesi a basso rischio. L'OMS ci ha elogiato e la maggior parte della stampa internazionale ha dichiarato che chi ha schernito l'Italia per le difficoltà iniziali

«Responsabilità» è, a mio avviso, la parola chiave per descrivere la validità e l'efficacia delle nostre strategie: responsabili le istituzioni, responsabili i cittadini e responsabile il personale sanitario, che, che, con un atteggiamento consapevole diffuso, hanno tutti deciso di rispettare le norme anticontagio. Abbiamo compreso meglio di altri che la nostra libertà si misura, non con il grado di anarchia, ma con la capacità di rispettare le minime regole di buon senso. Per una volta possiamo dircelo: siamo stati capaci, siamo stati bravi, in qualche modo. La scelta di un rilascio graduale del *lockdown*, di prolungare lo stato di emergenza, di continuare a mantenere l'obbligo delle mascherine è stata giusta - lo sappiamo - non è stato per niente facile. In questo senso dovremmo esprimere la nostra gratitudine al ministro Speranza, che ha tenuto duro nonostante pressioni enormi, rafforzate dalle prese di posizione irresponsabili di alcuni esperti. In Paesi come Francia, Spagna o Regno Unito, infatti, che a quelle pressioni hanno ceduto, stiamo assistendo a una seconda ondata che va assumendo contorni ancora più drammatici della prima, con uno scontro politico tra istituzioni che sta minando la coesione sociale. sociale. Guardiamoci allora attorno: la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio è la scelta più saggia e adeguata che si possa fare in questo momento. Ed è molto grave che, in una fase tanto drammatica e su un tema così importante, si sia fatta una insolente propaganda che nulla ha a che vedere con il senso di questa misura. Bisogna dire la verità: qui non si tratta di sospendere le libertà fondamentali o di attribuirsi dei pieni poteri, come qualcuno vuol far credere per fomentare lo scontro e trarne qualche vantaggio politico. La consapevolezza che lo stato di emergenza non si è concluso affatto consente al Governo e alla Protezione civile di usare procedure più snelle e veloci per emanare e fare applicare le misure necessarie per contenere un rischio epidemiologico maggiore. Si tratta dell'unico mezzo a disposizione per agire con tempistiche sufficientemente rapide, per monitorare in modo diffuso e costante, per aumentare quando occorre i posti in terapia intensiva, per dichiarare zone rosse in caso di focolai particolarmente preoccupanti, per garantire l'approvvigionamento del materiale legato al contenimento dell'emergenza e, oltre al versante sanitario, anche per non interrompere il lavoro, per mantenere le modalità di accesso allo *smart working*, rendendolo più facile per i genitori con figli piccoli, per attivare modalità più agili nell'assegnazione di appalti e coperture economiche speciali legati alla pandemia. Colleghi, un Paese serio si comporta così, perché senza regole non c'è libertà, lo ripeto: senza regole non c'è libertà. Questa è la fase più difficile. Siamo in un momento cruciale, dovremmo tutti remare nella stessa direzione, cercando di evitare gli errori commessi dagli altri Paesi che sono intervenuti quando era troppo tardi o quando i contagi erano altissimi. Il direttore generale dell'agenzia sanitaria della regione di Parigi ha dichiarato che il limite fissato è stato superato. Il nostro obiettivo - ed è una questione che dovrebbe riguardare tutti, dalla maggioranza all'opposizione - è attenerci alla prudenza, per evitare che i contagi raggiungano livelli altissimi e incontrollabili, e alla flessibilità verso le differenti situazioni specifiche a livello territoriale. I provvedimenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie servono a questo. L'imposizione delle mascherine anche all'aperto e il distanziamento sono misure necessarie per impedire contatti troppo stretti, per esempio all'uscita delle scuole o anche fuori dai locali pubblici. Dunque, una scelta di buonsenso. Per tutte le altre misure sono certa che la collaborazione tra le Regioni e il Governo consentirà di fare scelte che tengano insieme la necessità di tutelare la salute con la difesa dei redditi e del lavoro, oltre che della socialità, sia pure necessariamente ridotta e modificata. Non è semplice, non lo era ieri e non lo è oggi e, visto che nessuno vuole ripetere un *lockdown* che il nostro Paese non sarebbe in grado di reggere da alcun punto di vista, è indispensabile comportarsi tutti subito in modo serio, sostenendo ora le misure che ci aiuteranno ad evitare guai più seri in futuro. Servono sacrifici da parte di tutti affinché si dia reale attuazione alle misure di distanziamento sociale nei luoghi di assembramento dove ci sono maggiori rischi. Le regole ci sono, ora è necessario che siano fatte rispettare, tutto questo ci aiuterebbe a tenere aperte le scuole e - su questo credo siamo tutti d'accordo - tenere aperte le scuole è una priorità per tutti. Concludo proprio su questo aspetto: mi auguro che si lavori per ricostruire una nuova relazione organica e non episodica, come dichiarato dal ministro Speranza, tra il Servizio sanitario nazionale e il sistema scolastico, provando ad uniformare i protocolli di intervento delle ASL nei vari istituti ancora molto diversi tra loro, accelerando l'uso dei *test* rapidi che sono già stati acquisiti e che possono essere impiegati nei casi sospetti meno gravi. Colleghi, è evidente che di fronte a un'epidemia che colpisce tutto il mondo dobbiamo unire il Paese e non dividerlo. Per questo rivolgo un appello a tutti noi: l'intensificazione delle misure di sicurezza non diventi uno scontro di fazioni politiche, perché ne va del futuro del Paese.

lo scorso 14 luglio, quando in quest'Aula era venuto ad esporre i motivi per cui era necessaria una nuova proroga dello stato di emergenza fino a ottobre, avevamo già detto al Ministro che il nostro timore era quello che, senza soluzioni concrete in grado di contrastare efficacemente il virus,

per dirci quello che da giorni leggiamo sui giornali, ossia che l'aumento dei casi nel nostro Paese impone atteggiamenti di cautela e ulteriori restrizioni. Certo, serve cautela e responsabilità, ma leggere ad esempio che il Governo avrebbe intenzione di utilizzare l'esercito per controllare i cittadini che non indossano le mascherine all'aperto, sembra un po' una scelta azzardata o sbagliata. Noi siamo sempre stati per l'utilizzo dell'esercito nelle città, ma per la sicurezza dei cittadini. Questo utilizzo della paura e dell'incutere il terrore negli italiani sta portando veramente a un'enorme preoccupazione, direi anche all'esasperazione. Che cosa non ha funzionato in questi tre mesi nel concetto tanto caro a questo Governo delle tre «T», ossia tamponi, terapia, territorio? Avete valutato che forse il numero di tamponi per dichiarare guarite le persone inficia la capacità di testare i nuovi casi sospetti e i loro contatti? Mancano i tamponi, i tempi sono troppo lunghi. È chiaro il concetto per cui la *app* Immuni, che avrebbe dovuto dare una grande mano per implementare il tracciamento, non viene utilizzata? La gente ha paura di rimanere chiusa in casa a tempo indefinito perché l'ASL non provvede a fare i tamponi; passano otto o nove giorni. *(Applausi).* È stato giustamente ricordato tutto quello che riguardava la sierodiagnosi, ma sappiamo che è stata un fallimento la sieroprevalenza: su una previsione di 150.000 persone da testare, poi portate a 190.000, ne sono state testate dalla Croce Rossa soltanto 64.400. Le persone hanno rifiutato

al fondo affidato al commissario Arcuri. I test sono stati regalati dalle aziende e si è provveduto ad acquistare soltanto i reagenti, ma si è speso ulteriormente di più e la Croce Rossa ha speso ulteriori fondi delle donazioni. Sarebbe importante cercare di fare chiarezza ma questo stato dei numeri non si trova. Sappiamo che ci sono migliaia di persone, tra liberi professionisti e microimprenditori, con sintomi lievi che scelgono di non comunicarlo al proprio medico per paura di dover passare un lungo periodo a casa, e i test sierologici che dovevano essere usati per fare statistiche vengono rifiutati. rifiutati. Questi ulteriori mesi di proroga a cosa servono? Serviranno a migliorare questi sistemi? Con quali risorse? Perché non preparare al meglio i nostri ospedali e gli operatori sanitari utilizzando ad esempio i fondi del MES, che possono essere messi a disposizione subito? Io aspetto ancora una risposta ad una mia interrogazione di luglio che ho presentato perché tutto è fatto con estremo ritardo, la seconda ondata avanza, i cittadini sono nel panico in quanto temono la perdita del lavoro anche a causa dei figli, perché ogni settimana qualcuno resta a casa e non Certo che lo Stato e i cittadini devono collaborare attivamente e senza addossarsi le colpe reciprocamente, ma il caos dei numerosi provvedimenti non fa altro che creare confusione, mentre tutti avremmo bisogno di certezze

quanto ci facciamo i complimenti, quanto l'Europa e l'OMS ci dicono che siamo bravi»: sì, va bene, ma sono passati nove mesi. È stato un parto veramente lungo e difficile e direi che adesso vorremmo anche vedere il prodotto, il neonato.

Inoltre, chi pagherà una mascherina ogni quattro ore a 60 milioni di cittadini? Faremo nel prossimo decreto una norma che renda detraibile l'acquisto dei dispositivi di protezione? lei, signor Ministro, ha più volte detto che la drammatica situazione dei tagli alla sanità è finita e il sacrificio del Paese non andrà sprecato, proprio in ragione di una nuova programmazione che ci ha esposto con molta precisione in Commissione. Credo, però, che questa questa nuova stagione arriverà molto tardi, perché sul *recovery fund* si continua a litigare: le risorse pronte ci sarebbero fanno sì che forse ha ragione Sabino Cassese quando afferma che, più che davanti a una proroga dell'emergenza, siamo di fronte alla proroga dell'impotenza o alla proroga dell'incapacità.

ci indebitiamo di più», si aggiunge: ma non è che il *recovery fund* sono soldi che ci regalano, perché l'interesse da pagare è superiore a quello quasi nullo del MES. Non abbiamo più bisogno di assistenzialismo, del "Sussistan". Lei

Ci sono linee guida per i medici di base che rispondano al telefono e non facciano come nei mesi scorsi? Ci sono linee guida per l'assistenza territoriale? Come sono organizzate le ASL per avere i tamponi e l'esito del tampone in

sull'approvvigionamento dei farmaci antivirali utilizzati nei reparti Covid per curare i pazienti?

Signor Presidente, abbiamo ascoltato delle gran belle parole, dette anche molto bene, ma assolutamente lontane dalla realtà. neppure che stiate facendo tesoro di quanto vi abbiamo ripetutamente sottoposto in tutte le circostanze in cui ne abbiamo avuto occasione in materia di proroga dello stato di emergenza. Sono ormai nove mesi e anche un "parto difficile" dovrebbe giungere a conclusione, invece con la richiesta di proroga a tutto il mese di gennaio 2021 palesate che questi nove mesi sono trascorsi inutilmente, posto che non c'è alcuna evidenza di avere trasformato in procedure concrete e ordinarie quanto inizialmente avrebbe potuto essere giustificabile che venisse affrontato in regime di procedure straordinarie ed emergenziali.

l'indicazione del percorso da intraprendere: il piano di prevenzione, preparazione e contrasto dell'eventuale recrudescenza epidemica, nel quale avrebbero dovuto essere esplicitate e disciplinate le procedure per affrontare in modo tempestivo e appropriato tutte le azioni e gli interventi che sembrano essere indicati dal comitato tecnico-scientifico in quello che ha previsto come il peggior scenario da affrontare in caso di recrudescenza incontrollata. Scenario che avrebbe dovuto essere contemplato a luglio per essere evitato: sia per quanto riguarda i regolari approvvigionamenti (DPI), non solo le mascherine, sia sul versante dell'ottimale dotazione dei posti di terapia intensiva e semintensiva, sia per quanto

posto che continuate a prorogare lo stato di emergenza, delegando ad altri l'adempimento dei vostri compiti. Infatti, ad oggi, un italiano su tre non potrà essere vaccinato, con le dosi pianificate. Logica vorrebbe che, per recuperare in credibilità, trattandosi di un intervento emergenziale, lo smentiste in questa sede, con dati inoppugnabili, dando certezza del fatto che tutti gli italiani, in adesione consapevole, possano eccezionalmente fruire della vaccinazione antinfluenzale, quale livello essenziale di assistenza in emergenza, e non solo quindi per la profilassi della solita influenza stagionale, ma in quanto - come pare - blando antidoto anti-Covid. Anche di questo, volutamente e colpevolmente, vi siete dimenticati. Non c'è prevenzione senza controllo. Ecco perché abbiamo continuato a insistere e insistiamo sulla necessità di potenziare i controlli, sia nel pubblico che nel privato, e sulla necessità di ricondurre alla normalità alla normalità la regolazione degli atti di gestione dei fabbisogni di risorse umane e strumentali nella sanità post-prima emergenza, vale vale a dire superando la logica della gestione commissariale e della remissione al Comitato di decisioni che dovrebbero essere in capo Mi pare che ce ne sia abbastanza, ma vi aggiungo un'altra suggestione. La sinistra, che ha fatto della "demeritocrazia" un suo *mantra* dagli anni Settanta in poi, avendo il 18 politico e facendo sì che coloro che primeggiavano per profitto dovessero quasi vergognarsene e nascondere il fatto di essere i primi della classe nel segno dell'"uguaglianza al ribasso" anche remunerativa, ha prodotto tali e tanti di quei disastri, di cui oggi questo Governo è la prova provata della punta dell'*iceberg*. Anche quanto stiamo discutendo dimostra che non avete saputo o voluto trarre insegnamento dal periodo già vissuto obiettivamente a febbraio, marzo, aprile - un *unicum -* per mettere in campo quegli strumenti atti a fronteggiare con ordinarietà pericoli meno gravi. Non ci soffermeremo sulla capacità di risolvere i problemi, perché la vostra cifra è quella di trasferire sempre ad altri dell'operato, per cui non sapremo mai se si tratti di "debolezza" o di vera "incapacità". Il dramma è che siete al Governo senza una legittimazione, perché siete minoranza nel Paese, e se pensate il contrario allora non c'è nulla di meglio che andare ad elezioni perché la compressione sistematica delle garanzie costituzionali richiederebbe almeno una legittimazione da parte di una da parte di una consistente maggioranza; il vostro agire sarà pagato *obtorto collo* dalla totalità degli italiani di oggi e per le prossime generazioni:

abbiamo avuto riconoscimenti da testate giornalistiche, da economisti, ad esempio Paul Krugman ha detto che le nostre misure sono state tra le migliori scelte che si potevano operare; abbiamo avuto riconoscimenti Ghebreyesus, il direttore

al signor Vice Ministro, al comitato tecnico-scientifico con i suoi consigli e le sue raccomandazioni; grazie anche alla diligenza, intelligenza e civiltà del popolo italiano - questo non lo dobbiamo mai scordare assolutamente - che si è

i danni e le conseguenze negative di questa terribile pandemia. La pandemia purtroppo non è assolutamente terminata e fino a quando non avremo uno strumento terapeutico efficace quale può essere vaccino o un anticorpo monoclonale o qualsiasi altro farmaco in grado di distruggere il *virus,* laddove penetri dentro il nostro corpo, dobbiamo tenerlo lontano da noi, quindi dobbiamo continuare a osservare le regole di distanziamento di distanziamento fisico, di lavaggio delle mani e di uso della mascherina. Inoltre io esorto sempre i colleghi a scaricare l'*app* Immuni, che è di notevole importanza e utilità nel caso di tracciamento di possibili contagi. Gli ultimi dati sull'evoluzione della pandemia non sono sicuramente così allarmanti come nel resto nel resto del mondo, ma non sono neanche tanto rassicuranti perché la curva del contagio tende, seppur lentamente, a crescere; inoltre sono in parte cambiate le modalità del contagio, perché l'età mediana adesso si è spostata verso i

tipo intradomiciliare. Sono un po' diminuiti i focolai da *movida* e sono un po' aumentati quelli legati alle attività lavorative. Sono dati non allarmanti, che però ci inducono a tenere ancora sotto controllo, con grande senso di responsabilità, l'evolvere della pandemia. Ed è su questa strada che si deve continuare. Trovo quindi assolutamente ragionevole, comprensibile e giustificabile la proroga fino al 31 gennaio di queste misure, che fino ad ora ci hanno consentito di affrontare con efficacia l'epidemia. Vorrei ricordare, a quanti hanno parlato di libertà o di violata libertà, quello che ha detto

finiscono dove iniziano le libertà degli altri. Quindi usare cautela e prudenza e continuare con queste regole non mi pare assolutamente che possa privare gli italiani delle loro libertà, laddove si consente la continuazione in sicurezza delle attività formative, soprattutto delle attività scolastiche, e ovviamente anche delle attività lavorative. Non mi pare proprio che questa sia una limitazione delle nostre libertà. Per questo vi dicevo che a volte mi chiedo dove vivo, se in questo mondo e in questa Italia o in un'altra Italia disegnata non so per quale volontà politica. Accanto a queste misure a breve termine,

è malato. Lo abbiamo fatto ammalare e lo abbiamo fatto ammalare noi, lo ha fatto ammalare l'uomo. C'è un binomio indissolubile, un legame indissolubile tra ambiente e salute: se l'ambiente è malato, la nostra salute non si può considerare salute. Ricordo le parole di Papa Francesco: noi pensiamo di restare sani in un mondo malato. Non è così, perché più degradiamo l'ambiente

nella prossima programmazione per l'impegno delle risorse che verranno dal *recovery fund*, nella «missione salute»

proprio da medici ambientali (una figura professionale che in Italia manca) e da operatori ambientali. Ci sono i tecnici ambientali, ma manca la figura professionale del medico ambientale, cioè di quel medico che, formato specificamente (quindi occorrerebbe una scuola di specializzazione *ad hoc*), sia in grado di cogliere i segnali delle turbe qualitative del nostro ambiente di tradurle immediatamente in provvedimenti, perché questi segnali e queste alterazioni dell'ambiente, sia dell'ambiente sia dell'ambiente aereo che dell'ambiente terrestre o marino, inevitabilmente si ripercuotono sulla nostra salute. Questi medici dovrebbero avere quindi la funzione di sapere cogliere

avvengono invece interventi slegati, non coordinati, non omogenei tra di loro. A mio avviso e ad avviso di tanti colleghi, manca proprio questa figura.

al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

il Ministro per il suo intervento e per il lavoro che, con tutto il Governo, sta portando avanti nella gestione di questa emergenza sanitaria. Naturalmente, sono un po' sorpreso dagli interventi di alcuni colleghi in questo Senato, che hanno parlato di questioni che non stanno dentro il provvedimento che il Governo varerà questa sera. Si è parlato, ad esempio, di chiusura di attività economiche. Ebbene, vorrei ricordare che l'unica misura contenuta

Camera - è la previsione dell'obbligo delle mascherine all'aperto. Quindi, non c'è alcuna restrizione per quel che riguarda le attività economiche,

di gestione della crisi con il coinvolgimento diretto del Parlamento. Fino a qualche mese fa ricordo ai colleghi che il Consiglio dei ministri si riuniva e votava provvedimenti che comunicava successivamente alle Camere. Sottolineo in tal senso che è un successo di tutti noi, comprese le opposizioni, l'aver invece costruito un percorso diverso, tanto è vero che ieri si è riunito il Consiglio dei ministri ma non ha varato il provvedimento rinviandolo a questa sera a seguito della discussione delle Camere.

sono stati smentiti dagli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto da parte delle opposizioni. Un altro dato di fatto è stato negato dagli interventi che ho ascoltato: si è discusso come se il Paese non fosse ripartito. Noi per mesi, nei mesi del *lockdown* e nei mesi che lo hanno preceduto, ragionavamo tutti ragionavamo tutti sull'ipotesi della convivenza col virus: fino a quando il vaccino non sarà scoperto, in questo Paese bisognerà costruire le condizioni affinché vi sia una convivenza in alternativa alla chiusura totale. In

quella era la vera tragedia, non le mascherine all'aperto, Ministro. Vorrei che ci concentrassimo su questo e che capissimo come continuare a far funzionare il nostro sistema di protezione, sia individuale che collettivo, nell'organizzazione del nostro Paese, proprio per garantire che non ci sia più un *lockdown*. I più grandi *sponsor* del funzionamento del nostro sistema di protezione e della mancata diffusione del contagio sono proprio gli attori economici,

dice di stare attenti nella gestione dell'emergenza sanitaria, altrimenti si rischia di chiudere un'altra volta. Questo è il tema e su questo noi dobbiamo misurarci. Pertanto, l'invito che rivolgo ai colleghi dell'opposizione è a

mi rimbomba in testa e mi dà anche fastidio utilizzare la parola MES, perché l'abbiamo ripetuta talmente tante volte che, a questo punto, anche ascoltarla fa male;

rispetto al rischio di ripiombare in un'emergenza sanitaria straordinaria, dobbiamo anche tener conto delle risorse economiche che l'Europa, in maniera positiva, ci ha messo a disposizione per la gestione dell'emergenza sanitaria. Ciò che non comprendo è il motivo per cui questa maggioranza, ma anche molte forze d'opposizione, non tengano insieme le due questioni, se ci sono risorse destinate a quella misura, a maggior ragione quando vediamo

naturalmente mi riferisco a tutti quelli che non possono permettersi il costo di un tampone in un laboratorio privato, perché l'anomalia di questo Paese continua a essere presente: chi ha la disponibilità economica

e il contrario di tutto. Dopodiché, ci dice anche che abbiamo finalmente conquistato le libertà costituzionali. E meno male che abbiamo finalmente conquistato la normalità di un Parlamento che agisce nella pienezza dei suoi poteri e nel rispetto della divisione dei poteri!

chi più, chi meno - apprendiamo dalla stampa specializzata, dai giornali e dalle televisioni. È ovvio che stiamo parlando del tema del giorno e, quindi, tutti disponiamo della

Ministro, noi abbiamo adottato veramente misure restrittive, mentre altri Paesi europei non l'hanno fatto. Quella che oggi è la differenza fra noi e loro è esattamente questo: il *lockdown* che noi abbiamo adottato, la blindatura di tutte le attività e di tutti gli italiani nelle proprie abitazioni, non è stato fatto da nessun altro Paese e questa circostanza oggi vorrei dire vivaddio - torna utile in un diverso andamento della curva epidemiologica. Non poteva essere diversamente, perché oggi gli altri stanno facendo quello che noi abbiamo fatto a marzo, aprile e maggio. Era inevitabile che a Parigi chiudessero le *brasserie*, era assolutamente inevitabile che prima o poi lo facessero. Loro non l'hanno fatto

Rispetto a tutto questo, continuiamo a raccontarci, colleghi, una mezza favoletta: siamo stati bravi e tutti ci fanno i complimenti. Ebbene, ricordo al collega Pisani che tutti quelli che ci fanno i complimenti non votano non votano in Italia, ma votano quelli che in Italia giudicano quello che sta facendo il Governo. Allora, se voi siete sicuri, regalateci un Governo legittimo, portateci a votare un Governo legittimo e legittimato. Vedete, colleghi, uno dei motivi che soggiace al fallimento dell'indagine sierologica e anche al fallimento dell'*app* Immuni è che questo Governo non è riconosciuto dalla gente. La gente non si fida di quello che gli racconta questo Governo. È del tutto evidente che questo è il motivo per cui la *app* Immuni non viene scaricata; non è un complotto pluto-giudaico, è è che non si fidano dell'*app*, perché non siete capaci di raccontarla, oltre a spendere un mare di danaro più di quello che andava a speso. Rispetto a tutto questo oggi prorogare lo stato d'emergenza a un anno è un ossimoro, costituzionalmente parlando, perché lo stato d'emergenza c'è, è stato proclamato, anche a volte di oltre un anno, ma su circostanze precise, su pezzi di territorio circoscritti e non su tutto il territorio nazionale e su tematiche così general-generiche. Quindi, oggi non siamo assolutamente favorevoli a prorogare lo stato d'emergenza, che significa sostanzialmente tenere gli italiani in posizione prona. Gli italiani si devono rialzare, potendo fare affidamento su un Governo che li mette in sicurezza.

il Presidente del Consiglio, perché parliamo di prorogare lo stato d'emergenza e di continuare a condizionare le libertà costituzionali. Pertanto, se il Presidente del Consiglio trova la possibilità di andare ad Assisi e pronunciare la sua enciclica, andare a Venezia

quello che preferisce raccontare in televisione e senza contraddittorio. Deve venire qui a spiegarci quello che dobbiamo fare. cosa dobbiamo fare? Vede, Ministro, noi, a dieci mesi dall'emergenza, non ci sentiamo di continuare a condividere formalmente questi provvedimenti perché fino ad oggi abbiamo fatto leva solo su metà dei doveri che spettano a un Governo, la metà che attiene al richiamare i cittadini ai loro doveri. Abbiamo abbondato in questa metà,

È lo Stato che oggi deve rispondere; è lo Stato che deve riempire la sua metà di dovere, Ministro. Come lo deve fare? Adottando finalmente misure adeguate alla prevenzione, al contenimento e al contrasto dell'epidemia. È chiaro e noto a tutti cosa dobbiamo fare: adottare un piano pandemico, che non c'è. È la prima cosa da fare. Dobbiamo fare

Perché non possiamo farlo su tutto il territorio nazionale? Ci sono *test* rapidi adottabili in automedicazione. Diamoli ai medici di medicina generale e alle farmacie; chi vuole comprarsi il *test*, va in farmacia, lo compra e lo fa. Lei li ha citati, sono i *test* degli aeroporti. Dobbiamo fare i vaccini antinfluenzali; stiamo parlando, continuando a martellare i cittadini, della necessità di fare il vaccino antinfluenzale, addirittura l'antivirale, l'anti-herpes, e non ci sono i vaccini. Le farmacie denunciano che hanno 12 vaccini a farmacia. Cosa ci fa una farmacia con 12 vaccini? Spiegatemi cosa ci fa. Dobbiamo fare assunzioni in sanità. Abbiamo messo del danaro, abbiamo dato la possibilità alle Regioni di farlo, come abbiamo detto ieri,

ma anche di organizzazione e di turni di lavoro massacranti. Ministro, dobbiamo chiedere alla nostra comunità scientifica, a questo fantomatico Comitato tecnico-scientifico, quando la carica virale è capace di infettare,

non possiamo presumere che lui sia capace di infettare, dobbiamo saperlo con certezza. A nove mesi e oltre dall'insorgenza di A nove mesi e oltre dall'insorgenza di questo patogeno, possiamo pretendere che ci dicano quando un positivo senza sintomi non infetta e quindi probabilmente può continuare ad andare a lavorare e a esercitare la sua attività? dobbiamo aggiornare i protocolli alla mutazione del virus. Oggi, per esempio, c'è un paradosso; chiederò

e i medici di medicina generale sono il *front-office* del nostro Servizio sanitario nazionale. manifesta sintomi - e tra qualche giorno avremo tutta la sintomatologia legata alla sindrome influenzale - è evidente che chiama il suo medico di medicina generale. E il medico non può stare dall'altra parte del telefono perché non va a casa a visitare; non vanno E la gente è buttata lì, sperando che il buon Dio e le proprie difese immunitarie riescano a far superare loro una malattia che, magari, non è neanche diagnosticata, perché il tampone lo fanno dopo cinque-sei Tutto questo, signor Ministro, ci richiama a coprire quell'altra metà di responsabilità. Non chiediamo sempre agli altri, cioè ai cittadini, di essere responsabili, seri, attenti, accorti e prudenti. Cominciamo a farlo anche noi, a nove mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Abbiamo sulle spalle, tutti noi, 36.000 deceduti. deceduti. A questi 36.000 deceduti, alle loro famiglie, alle loro comunità abbiamo il dovere di dare una risposta di serietà e di competenza. Tutto questo va adottato e va adottato rapidamente. Volete fare la proroga dello stato di emergenza e la farete: la democrazia si basa sui numeri e, quindi, farete la proroga di questo stato di emergenza. Utilizzatelo, però, per adottare misure efficaci.

Colleghi, richiamo tutti al nostro senso di responsabilità, che riconosco essere generale in tutta l'Assemblea.

Presidente, colleghi, anch'io sono un po' colpito dagli interventi di questo dibattito. In genere non faccio mai polemiche, ma questa volta ne voglio fare una rispetto ad alcuni interventi. informare che la fiducia in questo Governo, proprio in relazione alla gestione del Covid-19, è stata dimostrata da come gli italiani hanno corrisposto alle indicazioni del Governo.

gli italiani hanno capito e hanno risposto positivamente. I dati dimostrano che la strategia portata avanti da questo Governo ha funzionato

Perché, colleghi, non riconoscere questo fatto? Non vuol mica dire che non ci siano problemi! Problemi ce ne sono e alcuni li solleverò anch'io. li solleverò anch'io. Su un passaggio così difficile, inedito e assolutamente impegnativo per la vita delle persone, però, importante che ci potessimo riconoscere in un risultato che è di tutti. Non è solo del Governo, ma di tutti, anche dell'opposizione e anche di quelli che dicevano

preparato, non avevamo le competenze. Quindi, è comprensibile che sia successo questo, ma quel risultato oggi ci consente di avere un dato profondamente diverso rispetto agli altri Paesi è un fatto molto importante, teniamocelo, valorizziamolo e impariamo dagli errori, come più volte ho cercato di dire.

diverso. Dopodiché, c'è un altro problema. Perché si arriva allo stato di emergenza? Su questo, in tempo di pace, secondo me, sarebbe giusto ragionare, perché tutto l'impianto legislativo di questo Paese rispetto alla funzione della Protezione civile, alle modalità di organizzazione, è legato a questa procedura, ma non è in discussione la libertà dei cittadini. Oggi non stiamo parlando di *lockdown*, non stiamo parlando di messa in discussione di questi elementi, stiamo cercando di trovare il modo migliore

e che nessuno voglia dire il contrario. Dopodiché, anch'io penso che bisogna fare qualche passo in avanti. In primo luogo, il Ministro ha detto giustamente che bisogna rafforzare il coordinamento con le Regioni. Qui, Ministro, c'è un problema: non si può una volta dire che le Regioni possono semplicemente e solo restringere le norme, la volta dopo che le possono anche ampliare e poi di nuovo che È arrivato il momento di stabilire con concretezza e chiarezza qual è il rapporto tra Stato e Regioni e chiarire che la gestione della pandemia deve essere veramente coordinata, perché, al di là di chi fa il primo della classe, con un'intervista o un *post*,

non ci può essere ulteriore discussione, almeno per quanto riguarda la presa di posizione del Governo e del Ministero. Ci sono poi delle scelte strategiche, lo abbiamo già detto, a partire dalla questione delle liste d'attesa; i colleghi l'hanno posta: giusto, giustissimo, anzi anch'io sono preoccupato.

è affrontata semplicemente con l'esternalizzazione e senza un progetto complessivo di riorganizzazione del sistema sanitario in questo senso e dei servizi, il rischio è che si vada ad una esternalizzazione strategica e definitiva; da questo punto di vista, sarebbe un problema.

Ministro, il suo Ministero e il Governo vi siete mossi benissimo sulla questione del vaccino, però è chiaro che c'è un problema più ampio nel rapporto tra le grandi imprese farmaceutiche, le forme le forme attraverso cui si definiscono i cosiddetti farmaci innovativi e la funzione di EMA.

è semplicemente perché il ragionamento sul valore aggiunto rispetto alla ricerca non faceva tornare i conti. Guardate che questo è un enorme problema. Negli Stati Uniti del presidente Trump - così evito di essere frainteso - si sta ragionando in modo su questo punto, e credo che l'Europa lo debba affrontare al più presto; diversamente, ci troveremo di fronte a delle sorprese rispetto al processo di innovazione strategica che ha la farmacologia nel mondo.

avrei sperato di iniziare questo mio intervento dicendo che qualche settimana fa, quando abbiamo affrontato questa stessa discussione, ci eravamo sbagliati; che le nostre previsioni, come qualcuno diceva in quest'Aula, erano eccessive e che, al di là della buona o della cattiva fede, sicuramente il quadro che prospettavamo era molto lontano dalla realtà. Questa mattina, al di là delle notizie apparse sulla stampa, le parole sobrie, rigorose, responsabili e serie del ministro Speranza, a nome di questo Governo, credo che inchiodino tutti noi a una difficile e amara verità. Lo dico rispondendo innanzitutto al senatore Romeo, che, tentando in qualche modo di fare un parallelo tra questa fase e quella del periodo più acuto del *lockdown*, ha che sostanzialmente, se paragoniamo il numero dei contagiati ai tamponi, non siamo poi in una fase così drammatica come invece viene descritta. Questo se ho interpretato bene le sue parole, Penso che le parole del ministro Speranza - e le abbiamo ascoltate tutti - abbiano in realtà detto ben altra verità, ovvero che sicuramente non siamo nella situazione di marzo-aprile - è sotto gli occhi di tutti - e ci auguriamo di non arrivarci di nuovo.

al sacrificio abnorme delle nostre strutture, del Servizio sanitario nazionale, dei nostri operatori, degli italiani che hanno risposto bene, quella curva aveva iniziato a piegarsi e a luglio e agosto avevamo raggiunto livelli di contagio e di occupazione dei posti in terapia intensiva sostanzialmente

Si sono adottati degli strumenti che, quando è stato drammaticamente e inevitabilmente necessario, hanno limitato la libertà dei cittadini.

non abdicazione di una funzione, perché c'è differenza tra rinunciare a esercitare una funzione e capire che è il momento di fare un passo non indietro, ma forse di lato,

davvero che da parte di tutti si riconoscesse che questi mesi non sono passati invano. Il Governo stesso ha utilizzato quei poteri, che gli sono stati dati

chiesto di capire qual è il piano, verso quale direzione stiamo andando e se il Governo ha costruito le condizioni per affrontare un'altra emergenza, qualora i numeri dovessero peggiorare peggiorare notevolmente e a tal punto da stressare il nostro Sistema sanitario nazionale. Ci si chiede quindi come ci siamo attrezzati. In questo caso la politica, che di solito viene accusata di essere la politica del "vorrei", "farò" e "dirò", ha portato dei numeri, che inchiodano tutti noi a delle verità, che non possiamo ignorare. Il ministro Speranza ci ha detto che siamo partiti con 5.000 posti di terapia intensiva, siamo ad 8.000 e arriveremo, grazie alle risorse stanziate

più necessaria sia sostanzialmente questa. Quindi abbiamo agito, e lo abbiamo fatto con rigore e senso di responsabilità. Ci accingiamo di nuovo a gestire l'attuale fase e chiediamo a tutti di partecipare e di fare

Forza Italia è stata la prima forza politica a denunciare il pericolo del Covid: fin fin dal 30 gennaio in quest'Aula, alla presenza del ministro Speranza, Forza Italia ha chiesto di affrontare molto sul serio questo pericolo, di adottare delle misure rispetto ai voli provenienti anche indirettamente dalla Cina, di prendere in esame l'uso delle mascherine. Parliamo del 30 gennaio, il giorno prima che il Governo approvasse lo stato d'emergenza. Tre giorni dopo, il 3 febbraio, in conseguenza dello stato d'emergenza,

la necessità di fermare o controllare strettamente i voli provenienti dalla Cina anche indirettamente, nel caso venissero da una zona particolarmente infetta; ora sappiamo che il mondo è cambiato da allora, ma l'epidemia viene da lì, e non da altrove; si era chiesto un controllo dei tantissimi bambini cinesi che tornavano nelle scuole, nel senso di sottoporli a quarantena: una misura che oggi sembrerebbe banale, ma che noi abbiamo chiesto il 3 febbraio. La senatrice Bernini, non da sola ma sostenuta anche da altri Capigruppo del centrodestra, venne ignorata in tali richieste.

In quella circostanza, di fronte al fioccare dei primi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo mantenuto un senso di grande responsabilità. Avendo noi per primi denunciato il pericolo, abbiamo coerentemente facilitato anche con le procedure parlamentari il compito del Governo di porre dei rimedi, di mettere mettere in atto delle misure per prevenire l'ulteriore espansione dell'epidemia, diventata nel frattempo pandemia, dando anche piena disponibilità all'Esecutivo attraverso la presentazione di una serie di proposte.

anche recentemente, quando abbiamo chiesto una vera moratoria, un vero rinvio di tante scadenze fiscali. *(Applausi)*. Abbiamo chiesto di non mandare milioni di cartelle esattoriali, tante delle quali sappiamo essere

da parte del Governo, che purtroppo abbiamo visto replicare proprio pochi minuti fa, quando il ministro Speranza, chiamato a rappresentare la posizione del Governo

ci torneremo; voi avete una posizione diversa ed è normale che respingiate la nostra richiesta di agire secondo quanto la Costituzione stabilisce, e cioè con un decreto-legge. Ma lasciamo stare; su questo ci torneremo. Noi abbiamo anche chiesto

Io non credo che lei, Ministro, sia contrario a predisporre un numero adeguato di vaccini antinfluenzali, ma il fatto di dire di "no", solo perché le firme erano quelle dei Capigruppo dell'opposizione, è esattamente l'opposto di avere

le linee guida relative all'isolamento delle classi e degli alunni in caso di sospetto contagio, al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità didattica. Può anche dire di "no", ma non sarebbe stato male fornire al riguardo una spiegazione. Devo dire che, con il degrado della vita vita parlamentare a cui abbiamo assistito in questa legislatura, dare spiegazioni è diventata una cosa più che rara, quasi stravagante, mentre invece il Parlamento serve proprio a questo, a dire davanti ai cittadini chi vuole fare qualche cosa e perché. A ciò dovrebbe servire il Parlamento; ma siccome qualcuno non ha capito bene a cosa serve, allora cerca di massacrare il Parlamento in tutti i modi. Noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio le misure di prevenzione e di prudenza, ma abbiamo anche ricordato i gravi costi che questo comporta. Ci sono i costi economici - e credo sia evidente a tutti

malattia, bisogna vedere di non concentrare gli sforzi solo su un aspetto. Come è stato detto anche da esponenti della maggioranza, ci sarà probabilmente un aumento di mortalità a causa di questa "monocultura" sanitaria. Bisogna affrontare le cose con il senso della realtà; ci vogliono trasparenza e chiarezza. Faccio l'esempio della promessa, data per certa, anzi addirittura approvata e messa per iscritto, di garantire un credito di imposta del 60 per cento per l'attività di sanificazione delle aziende. Benissimo. Tanti imprenditori, anche con piani importanti di grande impegno finanziario, sulla

Il Governo deve far fronte alla realtà usando i metodi previsti dalla Costituzione, che parla di decreti-legge, solo decreti-legge. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri servono per un'attività che sta al di sotto della normativa di legge; specialmente quando si limitano le libertà costituzionali è impensabile usare questo questo strumento, tanto più quando, per via dell'emergenza, si stabiliscono norme molto strane. Ricordo che ancora oggi non sappiamo quanto sono stati pagati i banchi nuovi, i famosi

Chiediamo al Governo serietà, senso della realtà, rispetto della Costituzione e dei cittadini che hanno fatto tanti sacrifici e hanno visto tanti morti. C'è bisogno di assoluto senso della realtà e - ripeto - rispetto per i cittadini: non promettere ciò che non si può mantenere e fare di tutto per risollevare il Paese. Noi lo facciamo ogni giorno con le nostre proposte, che chiediamo vengano ascoltate, altrimenti ve ne assumete voi la responsabilità, tanto più che usate strumenti non previsti dalla Costituzione.

concordiamo con le affermazioni del senatore Errani quando ci dice che questo è un risultato di tutti: è vero, collega, è un risultato di tutti, e lo diciamo con la stessa onestà intellettuale

Presidente, se cominciamo così non va bene. Lo ricordiamo anche a chi diceva «Bergamo non ti fermare!» per poi andare in vacanza a Formentera. Formentera. È un risultato anche di chi diceva «Milano non si arrende» e partecipava alla movida. Lo ricordiamo anche a chi diceva che i pazienti che non possono essere trattati sono lasciati morire, per poi essere smentito dal fratello medico. Lo ricordiamo per onestà intellettuale. Ministro, è dall'inizio della pandemia che vi stiamo invitando a una gestione più più condivisa e più oculata di quello che è lo stato d'emergenza. Nessuno in questo momento sta dicendo che lo stato d'emergenza non va bene. Diciamo semplicemente che lo stato di emergenza deve essere gestito in un modo diverso da come lo state voi gestendo. Vogliamo essere coinvolti. Chiediamo non che la minoranza sia coinvolta, ma che il Parlamento sia coinvolto, che è una cosa totalmente diversa. Ministro, la vostra gestione lascia alcune perplessità dal punto di vista sia tecnico che pratico. Dal punto di vista tecnico, Dal punto di vista tecnico, lo stato di emergenza è stato dichiarato in data 31 gennaio fino al 31 luglio; poi, venite qua e ci dite che è prorogato al 15 ottobre. Adesso ritornate a dirci che lo prorogate al 31 gennaio 2021: un anno di stato di emergenza, che va in senso totalmente contrario rispetto a quello che è venuto a dirci il Presidente del Consiglio in data 21 maggio. maggio. Il Presidente del Consiglio in data 21 maggio ci ha detto: «Non ci possiamo permettere di protrarre l'efficacia di misure così limitative per un periodo indefinito. Un ordinamento liberale e democratico non può tollerare una compressione dei diritti fondamentali». *(Applausi)*. Non l'ha detto Gian Marco Centinaio: l'ha detto Conte!

Confusione tra Stato ed enti locali: persino tra lo Stato e i Comuni c'era confusione, tanto che l'ANCI, in più di un'occasione, vi ha criticati nella gestione dei vostri provvedimenti. Imbarazzante, poi, Ministro, il rapporto tra il potere legislativo e il potere esecutivo, tra il Governo e il Parlamento, con il Parlamento come semplice ratificatore delle decisioni del Governo. Dobbiamo stare qui ad ascoltare e ad applaudire quello che decide il Governo, ma il potere legislativo è quello che rappresenta il popolo, è quello che è stato eletto dal popolo per decidere! *(Applausi)*. Non siete voi e i tecnici che ha pagato e strapagato il presidente Conte, ma siamo noi

libertà di circolazione, limitata; libertà di riunione, limitata; libertà religiosa, limitata; diritto all'istruzione, limitato; libertà di iniziativa economica, limitata; libertà personale, limitata. Queste limitazioni dovrebbero avere un rango di legge o di un atto avente forza di legge. È l'ABC della giurisprudenza. L'invito che le rivolgo, Ministro, e che rivolgo al presidente Conte, è di venire in Parlamento e di confrontarsi con il Parlamento. Ci sono i decreti, venite in Parlamento e ci confrontiamo. C'è poi tutto il punto di vista pratico. Le vostre decisioni, che prendete non si sa con chi - con noi non le prendete; magari le prendete con i vostri consulenti o con chi volete impattano sulla vita reale dei nostri cittadini, che le subiscono e le devono subire. Ministro, condividiamo la sua idea che ci voglia prudenza; ma la prudenza deve esserci anche nell'amministrare la cosa pubblica. Non si può amministrare la cosa pubblica come se fosse casa propria. Non state amministrando il vostro condominio: state amministrando il nostro Paese ed è una cosa totalmente diversa.

però, pensiamo anche che, se bisogna utilizzare l'Esercito, bisogna utilizzarlo per tutti, e non solamente per i pensionati che non utilizzano le mascherine, ma anche per chi arriva da fuori dai nostri confini e pensa di entrare a casa nostra e di vivere nel Paese del Bengodi.

alla sanità, state prevedendo un'eventuale crisi come quella che si è verificata l'inverno scorso? Non possiamo arrivare a dire che non eravamo preparati, avete avuto tempo per prepararvi, così come il ministro Azzolina ha avuto tempo durante l'estate di preparare l'accesso dei nostri figli nelle scuole.

Termino con due richieste.

Allora, o il presidente De Luca ha trovato la cura miracolosa e sta spendendo chissà che cosa, oppure i malati di Covid in Campania stanno negli alberghi a 5 stelle.

Vi dico subito che detta proroga è doverosa, giusta e necessaria e serve a tutelare e proteggere la salute degli italiani e, di conseguenza, a tutelare e proteggere la nostra economia, perché nessun rilancio dell'economia può essere raggiunto senza prima aver mantenuto in sicurezza la salute del popolo italiano. Questa scelta deriva dal senso di responsabilità con cui il Governo italiano ha gestito gli ultimi mesi difficilissimi, ma va anche ribadito che la proroga dello stato di emergenza - checché ne dica qualcheduno - non significa *lockdown*, perché questa falsità esiste solo per coloro che alla politica seria preferiscono la propaganda delle *fake news*. Sarebbe bastato leggere le norme per capire che non era così. Il decreto di proroga non chiudeva e non chiude in casa nessuno; anzi, mette in campo le condizioni proprio per evitare che ciò accada, grazie a strumenti più immediati ed efficaci di protezione dal contagio. Quindi, non servono allarmismi inutili. Non serve mettere in atto una strategia del terrore, tanto cara a qualche forza politica, così come non serve non serve sminuire la situazione che abbiamo vissuto e ci troviamo ancora a vivere. Anche questo è inaccettabile per tanti motivi. Da febbraio ad oggi abbiamo vissuto tante diverse situazioni. Siamo stati travolti da un vero e proprio *tsunami* che la mia Regione in particolare, la Lombardia, la Lombardia, ha subito in modo straziante. Abbiamo assistito a un aumento incredibile di contagi. Abbiamo assistito a un numero incredibile di decessi. Abbiamo visto mezzi militari lasciare Bergamo carichi di feretri. Abbiamo purtroppo assistito a una sequela di azioni da parte della Giunta regionale guidata dal centrodestra, che si sono tradotte in indagini *(Applausi)* e in inchieste giudiziarie che hanno inchieste giudiziarie che hanno profondamente colpito e turbato ogni lombardo. E, quando la situazione è iniziata lievemente a migliorare, oltre al danno, è arrivata la beffa, con i negazionisti e con chi qui in Senato ha addirittura organizzato un convegno rifiutandosi di indossare la mascherina: un insulto vero e proprio a tutti i medici e infermieri che ogni giorno lavorano in prima linea negli ospedali, alle persone che si sono ammalate, a chi ha perso la vita per il Covid, ai familiari e agli amici che hanno dovuto assistere da lontano allo strazio della malattia di qualcuno che amavano. Per fortuna in Italia a gestire la pandemia c'erano e ancora ci sono persone serie e responsabili e non i negazionisti o gli incerti del Covid, coloro che i giorni pari chiedevano di chiudere tutto e in quelli dispari di riaprire ogni cosa. Chiediamo però che d'ora in avanti ci siano più collaborazione e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, da parte di tutti. Ci attendono mesi importanti: impieghiamoli per uscire il prima possibile da questo periodo devastante. Abbiamo una base di partenza migliore di tanti altri Paesi al mondo; migliore perché siamo stati rigorosi nel predisporre le regole da seguire e gli italiani sono stati in rigorosi nel rispettarle. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Non è di certo il momento di mollare la presa oggi o di far scendere la tensione, perché è una sfida che si vince tutti insieme. Siamo tutti italiani e dobbiamo tutti remare nella stessa direzione, ma ciò avverrà se la politica tutta agirà in maniera responsabile. Lo chiediamo a coloro che negavano la pericolosità del Covid per andare incontro ai *desiderata* di una certa parte dell'elettorato che non condivideva le misure di prevenzione anti-pandemia. Lo chiediamo a chi non rispettava le regole di distanziamento sociale e di utilizzo delle mascherine, nonostante ricoprisse ruoli pubblici. *(Applausi)*. Lo chiediamo a chi attaccava la scelta di chiudere le discoteche per poi ritrovarsi esso stesso contagiato, insieme a molte altre persone. Lo chiediamo al Governo centrale e agli amministratori regionali e degli enti locali, affinché agiscano all'unisono, senza più polemiche e scaricabarili, perché ne abbiamo dovute sopportare davvero troppe. Lo chiediamo a chi addirittura ha parlato di un'Italia come fosse un "sussidistan", cioè un Paese fondato sui sussidi, ma non ci dimentichiamo che, dei cento miliardi e oltre destinati dal Governo in tutti i decreti emanati nell'arco del 2020, circa il 50 per cento è stato proprio destinato alle imprese. Allora guai a pensare che, se si danno soldi ai cittadini, sono sussidi e che, se invece li si danno alle imprese, sono strumenti di sviluppo e competitività. In questo senso, Presidente, voglio ricordare l'inutile e dannosa alzata di scudi contro il reddito di cittadinanza. Benedetto il reddito di cittadinanza, soprattutto in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto, dal quale non siamo ancora completamente usciti. chiediamo infine a chi per tutta l'estate ha attaccato il ministro dell'istruzione Azzolina che, a differenza di chi la contestava, ha lavorato ininterrottamente per permettere la regolare riapertura

È chiaro che il rischio zero non esisterà mai, ma è altrettanto chiaro che questo Governo ha messo in campo per la scuola molto di più di qualsiasi altro Paese europeo in termini di investimenti per la sicurezza. Abbiamo dovuto sentire stupidaggini sul plexiglass e altre *fake news* solo per screditare il lavoro che è stato fatto; continui attacchi a danno degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti. Noi oggi siamo l'unico Paese al mondo che manda tutti i giorni 11 milioni di mascherine chirurgiche *gratis* in 19.000 istituti scolastici italiani. È un dato oggettivo che non si riscontra in nessun altro Paese al mondo. La scuola è di tutti, signor Presidente, proprio come tutti hanno il diritto di essere curati. Sono principi della nostra Costituzione che in tanti e in troppi hanno dimenticato per il solo becero gusto di raccattare qualche voto che stavano perdendo. Gli italiani meritano uno Stato che sia all'altezza delle loro aspettative, che li protegga e li curi quando c'è bisogno; uno Stato dove non ci siano più cittadini di serie A e cittadini di serie B nel ricevere le cure sanitarie; dove i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari siano trattati come meritano. Non puoi chiamarli infatti eroi e poi assumerli come precari, come sta accadendo in Lombardia, dove è partito un bando da quasi 300 milioni di euro assegnato niente di meno che a tre colossi del lavoro interinale per la selezione di migliaia di infermieri e di operatori sanitari. Come non puoi elogiare gli ospedali di periferia, in prima linea nella lotta alla pandemia, come quelli delle Province di Lodi e di Cremona, e poi far chiudere interi reparti, se non addirittura ospedale interi. Tutto questo non deve più accadere. I soldi ora ci sono perché sulla sanità si è smesso di tagliare come è accaduto per troppo tempo in un passato anche recente. I soldi però devono essere impegnati molto meglio di prima. Vogliamo una sanità pubblica più forte e meglio radicata sul territorio. Sul punto stiamo lavorando e abbiamo lavorato. Non vogliamo una sanità pubblica fagocitata dalla sanità privata che si prende la metà dei soldi pubblici per gestirne solo la parte più remunerativa, quella che conviene - è questo sta accadendo ed è accaduto negli ultimi decenni in Lombardia - lasciando a quella pubblica le materie più complesse e meno remunerative. Tutto questo deve finire, come devono finire le porte girevoli tra la politica e i vertici dei colossi della sanità privata. Urla vendetta la nomina dell'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, all'interno dei vertici del più grande gruppo della sanità privata esistente in Lombardia. tutto questo conferma, una volta di più, che l'Italia deve dotarsi di una giusta, seria e rigorosa legge contro il conflitto di interessi. un altro traguardo che gli italiani attendono da decenni e che nessun altro partito ha mai realmente voluto. Ora però i tempi sono maturi anche per questo. Il tempo c'è, ma potremo portare a casa tutti questi risultati solo se continueremo a creare le condizioni affinché il Paese possa vivere, spostarsi e lavorare in sicurezza, facendolo però a pieno regime, invitando tutti a continuare a rispettare le misure di prevenzione e a difendersi con gli strumenti messi in campo da questo Governo, compresa l'*app* Immuni che ci aiuta a conoscere se siamo stati a contatto con persone positive al Covid. Iniziamo da qui, con un appello trasversale a scaricarla e a farla scaricare a tutti, anche a coloro che hanno avuto il coraggio di invitare le persone a non farlo. Iniziamo da qui, con questo segnale di unità nazionale e sono sicuro che gli italiani apprezzerebbero. Non ci dimentichiamo che la dal nostro Paese è stata lodata dalla comunità internazionale. L'ultima attestazione di stima è arrivata dall'Organizzazione mondiale della sanità, che non ha mai mancato di evidenziare come il modello italiano sia stato vincente nella gestione dell'emergenza. È proprio questo atteggiamento di precauzione e prevenzione che ha consentito al nostro Paese di gestire questo *coronavirus* meglio di tanti altri Paesi. Adesso che i casi di Covid-19 sono tornati ad aumentare in modo importante, prorogare lo stato di emergenza è davvero l'unico modo per continuare ad essere pronti in ogni momento; quella prontezza che tutti ci riconoscono; quella prontezza che, secondo alcuni studi, ci ha consentito di evitare decine di migliaia di morti. *(Applausi. La Presidente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

Dichiaro chiusa la votazione

sono venuti ad incontrare i dipendenti dell'aeroporto Canova di Treviso che, assieme a Venezia, costituiva in era *ante* Covid il terzo polo d'Italia dopo Roma e Milano è chiuso da marzo. I dipendenti sono in cassa integrazione, probabilmente fino a marzo dell'anno prossimo. Tutto il settore, quel piccolo, grande ecosistema economico che gravitava attorno all'aeroporto, è paralizzato. Molte aziende - mi riferisco al settore della ristorazione, dell'accoglienza turistica, perfino ai sistemi di trasporto locale, i taxi, ma anche alle aziende a servizio dell'aeroporto stesso - sono in crisi, a rischio chiusura. Da Treviso non arriva una richiesta di sussidio economico, l'appello non è per un salario minimo. Infatti, pende dinanzi al ministro dell'ambiente Costa la richiesta di un *masterplan* per l'ottimizzazione, l'ampliamento e la sostenibilità ambientale dell'aeroporto stesso, a capitale privato. In sostanza le società di gestione SAVE e AerTre hanno stanziato più di 50 milioni di euro per questo progetto vitale per rendere l'aeroporto redditivo nell'ipotesi che auspicabilmente questa crisi da Covid termini il prossimo anno. quindi, che rivolgo a nome di tanti cittadini di Treviso oggi in difficoltà non è una richiesta economica, ma è un appello affinché la maggioranza si trovi ad essere sensibile al grido di dolore di tanti che a Treviso stanno perdendo il proprio posto di lavoro e quindi chieda al ministro Costa di assentire e firmare l'autorizzazione, visto che comunque già due volte la commissione VIA si è espressa favorevolmente. Di conseguenza, non c'è un motivo per impedire l'ampliamento del nostro aeroporto, tanto più che, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, l'aeroporto è dal punto di vista logistico fondamentale. Non riusciamo a capire, a Treviso, perché si ignori la difficoltà, in un'epoca di crisi economica, per tante persone e tante famiglie che qui a Roma sembrano distanti, ma vi assicuro che tornare sul territorio e incontrare personalmente questa gente fa male. fa male. Chiedo quindi a questa maggioranza, che magari adesso è distratta (rivedrà il *video* forse più tardi) di agire nel senso già richiesto dal sindaco di Treviso Conte, da una mozione della maggioranza consiliare, ma perfino da esponenti del PD locale, che rimproverano alla Lega di essere passiva di essere passiva sull'ampliamento dell'aeroporto stesso. Prestate attenzione a questo problema e invitate il ministro Costa, cortesemente o meno cortesemente, a firmare l'autorizzazione per il *masterplan* nel nome del bene di tanti cittadini, alcuni dei quali in passato votavano anche il ramo sinistro di questo emiciclo. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli senatori, è bastato che ricominciasse a piovere per far riemergere il problema del dissesto idrogeologico, per far crollare i ponti, danneggiare strade e, fatto più grave, causare vittime. Però non possiamo attribuire la colpa solo al maltempo abbattutosi con particolare violenza, ma dobbiamo intervenire concretamente per impedire questo susseguirsi di tragedie e non lasciare che accada quello che invece si sta verificando per il ponte di Albiano Magra, crollato ad aprile 2020. era subito intervenuta nel *question time* con la ministra De Micheli per accelerare la nomina di un commissario straordinario incaricato di porre in essere i lavori in somma urgenza. Ciò è avvenuto con la nomina dell'allora presidente della Regione Toscana Rossi. Ma, a distanza di sei mesi dall'accaduto, nulla di fatto è stato realizzato e nel mese di settembre abbiamo proposto una nostra interrogazione urgente ai ministri De Micheli e Costa per evidenziare i gravi disagi e l'isolamento dei cittadini di tutta la zona interessata dal crollo del ponte, impediti finanche nell'accesso ai servizi sanitari di primo soccorso. Oggi, con la certezza che i Ministri interrogati intervengano con determinazione, sollecitiamo una particolare attenzione affinché comincino i lavori per la costruzione delle due rampe di accesso all'autostrada, per cui i sindaci del territorio stanno lavorando all'unisono e, in parallelo, si prosegua in maniera spedita con la costruzione definitiva del ponte. Concludo chiedendo che il Governo e anche il ministro Costa, di cui ho letto qualche intervista rilasciata, si ravvedano perché, proprio alla luce di una situazione che sta diventando ingestibile per i territori della nostra Italia, è necessario ripristinare al più presto la struttura tecnica di missione per il dissesto idrogeologico. avendo essa come compito quello di curare il coordinamento, la pianificazione e la gestione del rischio in Italia, avrebbe permesso un controllo più puntuale ed efficace dei fenomeni che, ad oggi, non si riescono a controllare.

Grazie, in ordine al maxiemendamento e a un rilievo della Ragioneria generale dello Stato su un emendamento, approvato all'unanimità in Commissione bilancio, che riguarda

prefigurato questa misura per le spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, cioè dopodomani, una manciata di settimane settimane nelle quali un cittadino, che magari sta aspettando da due-tre mesi il procedimento di ricostruzione, lo dovrebbe abbandonare per approcciarsi secondo gli interventi del *superbonus*, che dovrebbe realizzare in due o tre mesi. Capite bene che questa è una presa in giro, per cui rivolgo un accorato appello - vedo qui i rappresentanti del Governo - affinché in uno in uno dei prossimi provvedimenti, senz'altro nella legge di bilancio, si possa mettere mano a questa norma e si possa prorogarla per almeno due

nella disponibilità del Governo a prorogare questo termine. La Lega pungolerà attraverso interrogazioni ed emendamenti affinché questo possa essere messo nero su bianco. *(Applausi)*.

ma è un problema di non funzionamento del sistema del quale, se io non avessi avuto lo scrupolo di andare a chiedere lo stampato della votazione, non ci saremmo resi conto. Appellandomi alla sua sensibilità e a quella degli Uffici, ci tengo a evidenziare il problema; soprattutto, bisogna fare in modo che queste cose non capitino, perché non abbiamo automaticamente sempre